seguito e in connessione con la crisi e con quelle che sono dette risorse scarse e limitate. Su questo argomento tornerò successivamente.

sistema non è *in default*, allo sbando, ma è assolutamente ben controllato e seguito. Ripeto, la Commissione ha lavorato con impegno,

un importante e costruttivo incontro con il ministro dell'economia Tremonti. Vale la pena ricordare

egli ha definito una terra incognita: questa crisi ha scombinato tutti i sistemi e i rapporti, specialmente di tipo finanziario.

Il Ministro ci ha parlato dell'incertezza che serpeggia in tutti i Paesi industrializzati. Abbiamo però

di altre azioni importanti compiute, come il sostegno al settore produttivo, prevedendo l'accelerazione dei pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche per un circolante che manca. Abbiamo visto le azioni intraprese nei rinnovi contrattuali nel triennio 2010-2012; le modalità di contribuzione all'università, con un sistema dell'efficienza, dell'efficacia e anche un premio di risultato; la rimodulazione delle risorse dei Ministeri a favore di programmi prioritari,

che avrà il Paese, con la conseguente possibilità di agire in maniera più forte e concreta nel sostegno e nello sviluppo dell'economia.

forse più di tutto abbiamo analizzato lo spreco delle risorse, ed è nel momento di difficoltà che deve venire fuori la voglia di cambiamento e di rinnovamento.

vicino alla gente il punto di controllo e di comando, è far sì che i cittadini effettivamente controllino gli amministratori e questi si sentano responsabilizzati di fronte alla alla comunità che amministrano. Questo sistema Paese ha sempre diviso la responsabilità dal centro di potere. Così

È nella crisi che si fanno i grandi cambiamenti e i grandi passaggi: abbiamo la possibilità di farlo, il Paese lo chiede, e lo dobbiamo fare. *(Applausi

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ormai il quadro sullo stato del comparto agricolo è noto. Ogni giorno ne viene denunciata l'emergenza: lo fanno le associazioni agricole e gli stessi produttori in mobilitazioni, presidi, manifestazioni, al Sud come al Nord, i piccoli come i grandi produttori. I dati e le analisi ormai coincidono: le imprese sono strette tra un aumento dei costi e un calo delle quotazioni all'origine che fa crollare la redditività delle aziende. I prezzi all'origine si sono ridotti ulteriormente: del 20 per cento i cereali, del 22 per cento la frutta, quasi del 20 per cento i vini. Sappiamo del crollo del prezzo del latte in tutta Europa, abbiamo visto le immagini. Sappiamo della zootecnia, il cui arretramento è ormai pluriennale. In sostanza, Presidente, se il settore agroalimentare nel suo complesso può registrare dati di tenuta, la situazione è gravissima come non è mai stata, come nessuno ricorda per i produttori: non tutti i soggetti della filiera, ma l'anello più debole, il più critico, i produttori, il cui reddito dal 2000 ad oggi è sceso del 20 Ed è un indebolimento che, dobbiamo saperlo, non è solo economico. Sta avvenendo una trasformazione preoccupante: il produttore sta perdendo peso e autonomia nella capacità di governo del proprio prodotto nel percorso che va dal campo allo scaffale. Lungo la catena del valore dal produttore al consumatore chi detiene più marginalità di reddito è la rete della trasformazione, sono i soggetti che posseggono le reti della commercializzazione. Il produttore è l'anello più vulnerabile: sempre meno ha potere di contrattazione con la grande distribuzione, sempre meno - dunque - intraprende, sempre più lavora "per conto". E se non avessi timore di banalizzare, parlerei di una nuova forma di mezzadria del nuovo secolo che avanza, perché questa è la portata della debolezza che sta emergendo tra i produttori. Se non intravediamo questo rischio abbiamo anche noi, come classe politica, una grande responsabilità. Per tale motivo dico che dobbiamo prendere coscienza che siamo di fronte ad una crisi complessa, perché è la somma di più fattori: è debolezza strutturale, che non è di oggi; sono politiche europee, che assistono sempre meno; c'è un crisi delle materie prime, che si porta dietro le relative speculazioni; c'è l'effetto della crisi finanziaria. Inoltre, è un fenomeno che riguarda tutta Europa e non solo noi. Qui, allora, non si tratta di improvvisare, di misure estemporanee, di rassicurazioni e *spot* mediatici: qui c'è bisogno di un piano di grande responsabilità che affronti non solo la congiuntura, ma il medio e lungo periodo, la prospettiva di questo settore, che sappia mettere insieme l'emergenza, che vuol dire far fronte subito all'emergenza liquidità delle aziende per sostenere il peso dei mutui contratti in questi anni per alleggerire i costi del lavoro. Un piano che coraggiosamente punti ad un rafforzamento del sistema produttivo agricolo, che lo spinga all'aggregazione, al fare insieme, ad ottimizzare i costi e a correggere anche inefficienze che lo stesso sistema si porta dietro. Un progetto complessivo: lo diciamo e continuiamo a sostenerlo con forza come Gruppo del PD. Abbiamo presentato interpellanze, mozioni e un disegno di legge articolato che contiene i pezzi di un disegno a medio termine, basato proprio sull'emergenza e sul rilancio insieme. E non è una proposta teorica di un Gruppo di opposizione. Lo sta già facendo la Francia, e così lo ha presentato il presidente Sarkozy nei giorni scorsi: un piano senza precedenti di sostegno eccezionale al settore agroalimentare di 1.650 milioni di euro, con misure immediate per il credito e, insieme, misure per l'ammodernamento, un piano che guardi al futuro. futuro. Al contrario, il Governo italiano, come sempre, fa annunci. Annuncia nel DPEF l'esigenza, per quanto riguarda il settore agricolo, di rafforzare la competitività delle imprese, la stabilizzazione della pressione previdenziale, il sostegno agli investimenti, la crescita dimensionale delle aziende, una prospettiva pluriennale di finanziamenti e degli strumenti assicurativi. Chi più ne ha più ne metta. Poi, nella legge finanziaria nulla: l'unica norma agricola è un "salvaconti" sulle pensioni agricole e una interpretazione che eviti un appesantimento sui conti pubblici. era attesa dal mondo agricolo, ora, una presa in carico del settore. Erano attese almeno misure di emergenza come le agevolazioni contributive, l'estensione della "Tremonti-*ter*" sulla defiscalizzazione degli utili reinvestiti per gli investimenti in macchinari e attrezzature agricole, che hanno visto una contrazione di oltre il 20 Soprattutto, era attesa un risposta su quella che è diventata un chimera: il Fondo di solidarietà nazionale, pluriannunciato dallo stesso Presidente del Consiglio, promesso ogni volta un po' più in là. Intanto gli scoperti dei finanziamenti hanno messo in grande difficoltà i consorzi e gli imprenditori. Sappiamo di questa micromanovra agricola contenuta nel disegno di legge recante "Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare", in discussione alla Camera. Un provvedimento parallelo che cerca di tamponare che prevede un terzo delle risorse per il Fondo di solidarietà, una microproroga (si parla di mesi) delle agevolazioni contributive ed altre misure sul credito, il tutto con una previsione di copertura finanziaria derivante dai capitoli delle bioenergie, ovvero una coperta che, alla bisogna, si sposta: copre da un lato e scopre dall'altro. Siamo ben lontani da un programma di prospettiva, dall'occhio lungo di un governo politico dei fenomeni. Siamo ai tatticismi di giornata per coprire una manovra che abbandona a sé il settore e non se ne occupa. Ci dica finalmente cosa vuole fare questo Governo sull'agricoltura. Ci dica qual è il percorso, quali gli obiettivi, per arrivare dove. Siamo disposti a ragionare di tappe, ma su un programma, su un disegno articolato. Per i giochi delle tre carte, per gli *spot* e gli annunci il tempo è scaduto: la gravità della situazione non li permette più.

discute seriamente al proprio interno delle linee di politica economica. Non lo dico polemicamente, ma in termini assolutamente positivi perché lo sta facendo con gli strumenti che le istituzioni mettono a disposizione: attraverso emendamenti e, quindi, aprendo un dibattito che non potrà che essere positivo. Invece, la vera novità negativa - se di novità si può parlare - è che c'è, a questo punto del dibattito, il forte sospetto che tale apertura di discussione sulla linea economica della maggioranza stia ormai sfociando in un

Lo dico in termini di esperienza diretta, perché anche nella passata legislatura, quando al Governo c'era pure il mio partito, si sono fatte manovre dettate dalla contingenza, ma,

Voglio fare due premesse di ordine generale che sono necessarie perché non si ingenerino equivoci su quanto sto dicendo. Personalmente sono, come sicuramente tutto il PD, per il rigore dei conti: su questo non devono essere ingenerati dubbi. Sul rigore dei conti nella passata legislatura qualche prezzo il PD lo ha pagato perché il rigore dei conti non è esattamente popolare in questo Paese. Devo anche dire che ho apprezzato - l'ho detto in quest'Aula - la gestione oculata della crisi che un anno fa fece il Ministro dell'economia. Nel momento in cui la genesi e l'evoluzione della crisi economica erano da sfera di cristallo; il Ministro è rimasto immobile, perché non si imbastiscono politiche economiche sulle congetture. E fino a quel punto ho convenuto. passato un anno: se quella politica era comprensibile e adatta nel momento iniziale della crisi - una crisi dalla genesi e dagli sviluppi del tutto incerti - oggi questo è puro immobilismo.

per una crisi che ormai ha dei numeri totalmente definiti. Non siamo più sul piano delle congetture, ma su quello dei dati reali che il Governo ci ha fornito. E il Governo nei suoi documenti ci sta dicendo che

assolutamente asfittico: la previsione di una crescita del PIL dello 0,7 per cento fa tremare le vene ai polsi, se a questo aggiungiamo l'altro dato - anche questo incontrovertibile - fornito dalle istituzioni ufficiali e dai documenti del Governo, di un debito pubblico che è al 118 per cento già a fine del 2009. Queste non sono più

A meno che, ovviamente, non si sia anche su questo problema fermi alla puntata precedente. Ho infatti la sgradevole impressione che proprio la lunghezza delle nostre determinazioni sulla materia economica ci porti sempre a discutere della puntata precedente. precedente. Vorrei che la maggioranza prendesse in considerazione proprio la necessità di intervenire, certamente sull'IRAP, che è un problema che da tempo viene posto, e di intervenire nei termini strutturali che ho testé ricordato,

inutile tagliare l'IRAP se oggi tutte le piccole aziende ci stanno dicendo che non hanno ordini e, quindi, hanno un problema di fatturato. Il fatturato - come ci stanno dimostrando in termini molto chiari - si produce attraverso altri stimoli. La rottamazione ha funzionato

di un lavoro sicuramente pesante e impopolare, ma che non può essere rimandato, perché ogni problema messo sotto il tappeto riemerge drasticamente - e peggiorato - se non viene affrontato. Guardate, colleghi, che uno spazio c'era: gli emendamenti presentati dalla maggioranza, per molti versi, sono simili ai nostri; quindi c'era una possibilità di aprire su questo punto un dialogo serio. Ora, invece, abbiamo sostanzialmente davanti due strade:

studiamo una versione condivisa. Il conto da pagare alla crisi è altissimo e le debolezze strutturali del Paese sono enormi: assunti questi principi e avuta da parte del PD una serie di emendamenti sicuramente aperti al confronto

*(LNP)*. Signor Presidente, colleghi senatori, questa finanziaria che stiamo discutendo è sicuramente un nuovo tipo di manovra: una finanziaria snella, virtuosa, che cerca il più possibile di affrontare il tema della razionalizzazione della spesa, piuttosto che adottare la solita vecchia modalità dei finanziamenti a pioggia, che purtroppo ha contraddistinto il passato anche recente.

molti di questi vadano a buon fine. Parliamo di cose tecniche e forse anche un po' assurde ed anacronistiche. Stiamo chiedendo l'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili (la famosa ICI), che purtroppo ad oggi alcuni Comuni stanno applicando per gli impianti fotovoltaici messi a terra. Mi sembra un po' assurdo mettere una tassa sulle energie alternative. Abbiamo presentato inoltre alcuni emendamenti che riguardano la possibilità di aumentare i benefici per quanto riguarda lo scambio di energia per gli impianti fotovoltaici delle amministrazioni pubbliche. Oggi possono beneficiarne i Comuni fino a 20.000 abitanti; noi chiediamo che questo beneficio possa essere esteso a

in maniera climatica. Sappiamo benissimo che le ore di sole al Nord sono inferiori a quelle del Sud; quindi sarebbe forse giusto, da parte di questo Governo, rivedere i contributi del conto energia almeno nella loro durata, per far sì che possano essere incentivati di più gli impianti fotovoltaici al Nord, dove forse sono anche più necessari, visto il grande, forte e costante bisogno di energia. Questa finanziaria

Era la triste notte del 6 aprile quando una scossa di circa 6‑7 gradi della scala Richter ha devastato quella zona. Credo che sia giusto e doveroso fare

di euro, più altri 7 miliardi per la ricostruzione, compresa la messa in opera di 5.000 case prefabbricate, antisismiche ed ecocompatibili, per affrontare nell'immediato le esigenze di 13.000-15.000 sfollati che hanno avuto la casa interamente distrutta. Entrando nel dettaglio, il Governo ha erogato 150.000 euro subito a chi avesse provveduto da sé alla ricostruzione della propria casa ed ha erogato 80.000 euro se c'erano da riparare delle lesioni. Alla Regione Abruzzo sono arrivati 220 milioni di euro,

per quanto riguarda le imprese sono stati previsti vari indennizzi. Sono stati sospesi i pagamenti tributari e previdenziali, nonché i pagamenti degli affitti e delle rate del mutuo.

nel periodo di tempo che va dal 2009 al 2033 saranno investiti ben 6.924 milioni di euro. Una cifra che serve; se è stata data, significa che ce n'era bisogno. Ricordo a tutti che la Lega Nord è prontamente intervenuta,

di altruismo, inviando uomini e risorse là dove ve ne è stata necessità ed utilizzando il volontariato o tramite le istituzioni.

Il nostro territorio ha dato e sta ancora dando molto, forse anche troppo, considerati i risultati finora ottenuti. Siamo in attesa che con il federalismo fiscale e magari con i decreti attuativi si riesca quanto prima a lasciare un po' più di risorse nel nostro territorio.

condivisione anche negli altri Gruppi, non solo negli alleati del Popolo della Libertà, ma anche nel Partito Democratico, nell'Italia dei Valori e nell'UDC. Credo sia impossibile non accogliere tale emendamento, con quello spirito di responsabilità con quella solidarietà che contraddistingue noi, come movimento della Lega Nord, ma che, a mio avviso, contraddistinguerà anche tutti i politici di buon senso presenti in questa Aula.

ponendo una domanda fondamentale, soprattutto sulle tabelle riguardanti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La domanda è se si voglia fare una politica delle emergenze, una politica di sistema

Affrontare una riflessione sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il 2010 è, da un lato, semplice perché i dati parlano da sé e sui tagli non c'è questione; dall'altro, è difficile, perché sfugge il senso delle scelte soprattutto nei settori strategici (potremmo fare un lungo discorso sulla *green economy*, per esempio, sullo sviluppo sostenibile e sulla ricerca). sfugge anche il senso delle scelte in settori di vitale importanza per il Paese (dove il termine vitale assume una pregnanza particolare) come la conservazione dell'assetto idrogeologico del nostro territorio. Non si capisce cosa sia accaduto su questi capitoli di spesa

e in considerazione dei durissimi risvolti che la crisi ha avuto ed ha in campo occupazionale, la consapevolezza che un'economia legata a produzioni e consumi ambientalmente positivi e vantaggiosi sia non solo valida in sé sia anche uno dei terreni più fertili per sviluppare politiche economiche in contrasto con la crisi. Così, in numerosi piani di contrasto alla crisi dei Governi dei maggiori Paesi industrializzati, Paesi industrializzati, la *green economy* è diventata una scelta importante e consistenti investimenti e varie forme di incentivazione sono risultati centrali. Basti pensare al campo dell'efficienza energetica, allo sviluppo delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile. Secondo studi recenti, il peso percentuale di tali misure nei piani destinati a far ripartire le economie nazionali

Da ultima arriva l'Italia, con una percentuale dell'1,2 per cento delle risorse aggiuntive impegnate in tale campo. I dati, come dicevo, si commentano da sé. Tra l'altro, la *green economy* costituirebbe, se pensiamo al settore dell'efficienza energetica, un punto di incontro tra due esigenze altrettanto importanti: rilanciare gli investimenti e avviare decisamente politiche ambientali virtuose con conseguenze benefiche sulla qualità dell'ambiente, sulla riduzione dei costi energetici per imprese e famiglie, sulla dipendenza dei sistemi energetici da fonti fossili (che per l'Italia rappresenta una delle questioni centrali per le importazioni e per i costi generati al sistema) e, ancora, con conseguenze benefiche sull'innovazione tecnologica e sulla riduzione in atmosfera di emissioni dannose. Di tutto questo, è del tutto evidente la pressoché totale la pressoché totale mancanza di consapevolezza sia sotto il profilo ambientale sia sotto il profilo economico, a breve termine e a lungo termine. Persino misure minime condivise ed apprezzate nel Paese, come gli incentivi alle ristrutturazioni finalizzate al risparmio energetico, scompaiono con tutto quello che si portavano con sé in termini di consapevolezza ambientale per i cittadini e di motore economico. Intanto, Francia e Regno Unito varano leggi per cui, a breve, tutte le nuove costruzioni dovranno produrre persino più energia di quella che consumano.Siamo di fronte ad un vero e proprio arretramento delle politiche per l'efficienza energetica e questo non fa ben sperare circa il ruolo che l'Italia avrà nei prossimi appuntamenti internazionali, *in primis* la Conferenza sul clima di Copenhagen. Del resto, è massacrato persino lo stanziamento su ricerca e innovazione che, a fronte di un assestato del 2009 di 114,2 milioni di euro, si ferma, per il 2010, ad una previsione di 91,3 milioni di euro, con una riduzione di 22,9 milioni. Ma torniamo al cuore delle politiche ambientali del Governo, quelle previste - usiamo il riferimento al cosiddetto ecobilancio - per la missione 18, che si occupa dello sviluppo sostenibile e della tutela del territorio dell'ambiente. Se guardiamo ai totali delle previsioni non possiamo che essere sconcertati. Restano 595,9 milioni di euro, a fronte di una riduzione di 516,6 milioni di euro rispetto all'assestamento del 2009. Ecco, chiedo al collega che mi ha preceduto come sia possibile ragionare su nuove emergenze, a fronte di quello che è accaduto in questa missione. Qualcuno potrebbe pensare a virtuosi tagli di spesa improduttiva e, date le ripetute e roboanti dichiarazioni di qualche Ministro sul funzionamento della macchina statale, lasciarsi attrarre da tale idea. Ma andando nel dettaglio viene, invece, da chiedersi quale Paese conoscano i Ministri e, in particolare, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il primo punto riguarda la conservazione dell'assetto idrogeologico. È di tutta evidenza che questa spesa non possa dirsi improduttiva in un Paese che ha ferite recenti come il terremoto d'Abruzzo, con i suoi morti, e come il disastro di Messina, o come le più piccole ma devastanti alluvioni che qua e là costellano la vita di centri operosi e vitali, come è stato ricordato poc'anzi. E non è solo un problema ambientale, ma troppo spesso di vite umane spezzate e di luoghi che da amici diventano nemici e ostili per coloro che li abitano. Il dissesto idrogeologico e il rischio sismico rischiano di diventare pericolose costanti della vita del Paese. Ebbene, a fronte di una previsione di assestamento del 2009 di 271,7 milioni di euro, si passa ad una previsione per il 2010 di 120,8 milioni di euro. E non si parla qui di interventi eccezionali che - è vero - sono previsti nei documenti al nostro esame, bensì di conservazione dell'assetto idrogeologico che già lo scorso anno aveva registrato riduzioni di stanziamento. Il resto della missione 18 è un bollettino di guerra: meno 75,5 milioni di euro per la previsione e riduzione dell'inquinamento; meno 196 milioni di euro per lo sviluppo sostenibile; meno 17,4 milioni di euro per la tutela e la conservazione della biodiversità; riduzioni anche nel campo della vigilanza e repressioni in materia ambientale e, *dulcis in fundo,* meno 79,4 milioni di euro per il trattamento dei rifiuti, le bonifiche e le risorse idriche. Non credo che la lista che ho appena fatto appartenga alle spese superflue. Non sono più finanziati investimenti importanti per la conservazione dell'assetto idrogeologico e il grosso della riduzione in tale materia riguarda i piani strategici nazionali e l'intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico per favorire forme di adattamento dei territori da attuare d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati. Allora, ci diciamo che stiamo facendo una previsione seria sul rischio idrogeologico in questo Paese? È davvero difficile, dopo un anno come il 2009, capire questa scelta. Analoghe riflessioni potrebbero essere fatte sulla riduzione di risorse per lo sviluppo sostenibile. Che ne è del fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra? meno 196 milioni di euro riguardano essenzialmente questo fondo)? Che ne sarà della posizione e del ruolo dell'Italia

Sono presenti e assistono alla nostra discussione, in occasione della loro visita al Senato, gli studenti del Liceo scientifico della Scuola Pontificia «Pio IX» di Roma. A loro e ai loro insegnanti rivolgiamo il nostro saluto e gli auguri per la loro attività di studio.

Scelgo di parlare principalmente di tale settore, perché mentre tutti gli operatori aspettavano ristoro dal provvedimento in discussione, non solo esso non porta un solo euro in più rispetto all'anno scorso ma al contrario opera ancora tagli incondizionati e completamente slegati da qualsivoglia programma di riordino del settore. Paghiamo ancora, e forse pagheremo per molto, gli effetti del famigerato decreto-legge n. 112 del 2008, che tanto danno ha fatto e sta continuando a fare a settori vitali dello Stato: ad esempio, per citarne uno, alla scuola, Badate bene, colleghi, dico "tanti danni ha fatto", non perché l'Italia dei Valori sia semplicemente a difesa del carrozzone pubblico e quindi contraria ad ogni tipo di taglio di fondi. Riteniamo che sicuramente si dovessero operare dei tagli in determinati settori della pubblica amministrazione che funzionano male. Tuttavia, pensiamo che i tagli andassero operati con un programma di rivisitazione di interi settori da riformare e non solo da ridimensionare. L'esempio emblematico è la Difesa, un settore che ha subito tagli anche del 40 per cento delle dotazioni. Mi preme sottolineare che il settore più penalizzato dal decremento di risorse è quello delle spese per il personale militare e civile (219 milioni di euro in meno). Leggo che tale decremento è «dovuto sostanzialmente a una riduzione dei volumi di forza di circa 10.289 unità rispetto al 2009». Pertanto, i fondi destinati alla professionalizzazione delle Forze armate, che già quest'anno avevano subito un grave taglio del 7 per cento, arriverebbero nel 2010 a diminuire di un pesantissimo 40 per cento, andando ad esasperare ulteriormente il problema del precariato nelle Forze armate e provocando la delusione di altri giovani che, nonostante l'impegno profuso nella formazione militare, non vedranno concretizzarsi la possibilità di inserimento. 127 milioni di euro vengono sottratti alle spese di esercizio. Le conseguenze di ciò sono evidenziate nella Nota preliminare, che recita testualmente che in tali condizioni «le aree afferenti il mantenimento e la manutenzione generale dei mezzi ed equipaggiamenti, dei servizi generali, delle strutture e di ripianamento delle scorte, permangono e anzi accentuano la loro condizione di forte sottofinanziamento e sono destinate a peggiorare vertiginosamente». compromettono la capacità e la prontezza operativa dello strumento militare. È in queste condizioni che continueremo a far affrontare ai nostri soldati le diverse missioni all'estero in cui il nostro Paese è impegnato a livello internazionale, come quella in Afghanistan? Si tratta di tutti quei militari, compresi i carabinieri, che pattugliano il nostro territorio, e dei nostri soldati che proprio in questi giorni ci preoccupiamo di onorare istituendo il Giorno della memoria dei caduti nelle missioni internazionali di pace; così come ci preoccupiamo ogni sei mesi di coprire il loro costo quando li mandiamo all'estero. Di questo passo, i nostri militari non potranno più pattugliare il territorio, perché non ci sarà più benzina per le loro macchine, non potranno più volare per l'assenza di risorse per il mantenimento in efficienza degli aerei. Insomma, non potranno più esercitarsi sui mezzi con i quali, qualche mese dopo, andranno in missioni all'estero! Tali elementi non fanno che comprovare un *trend* ulteriormente peggiorativo dello stato già troppo problematico in cui versano le nostre Forze armate e tutto l'apparato tecnico-amministrativo del Ministero. In questo quadro delle cose non si riesce neppure a sperare che durante il prossimo anno il processo di ristrutturazione indispensabile alla Difesa possa cominciare a produrre i suoi effetti. C'è però dell'altro. Ci sono responsabilità specifiche del Governo, e voglio sperare non della maggioranza, che fa ancora in tempo a ravvedersi, nel momento in cui, come è accaduto in Commissione bilancio durante l'esame di questo provvedimento, di questo provvedimento, richiede e approva emendamenti che addirittura prevedono l'istituzione di società, cosiddette *in house*, a cui il Ministero della difesa dovrà subappaltare le importantissime competenze in materia di acquisti di ogni genere e vendite dei propri marchi. Mi rivolgo al Governo e alla maggioranza che lo sostiene, Presidente. Che bisogno c'è oggi di approvare l'istituzione della società «Difesa Servizi Spa» tramite un emendamento alla legge finanziaria? Perché ci si presta a giochetti di questo tipo, approvando nella notte, nel silenzio di una Commissione composta da poche persone, un testo riguardante un ente cui lo stesso Governo ha pensato bene di dedicare un disegno di legge apposito? Perché, colleghi della maggioranza, avete votato a favore di questo emendamento in Commissione bilancio? Non siete forse certi della bontà del lavoro che i vostri stessi colleghi di maggioranza svolgono in Commissione difesa, peraltro guidati egregiamente dal presidente Cantoni? L'Italia dei Valori non può pensare di prestare il fianco a operazioni del genere. Noi ci opponiamo, e avremmo voluto avere la possibilità di presentare emendamenti soppressivi dei commi in questione. Ci opponiamo, Presidente, per il modo con il quale procedono i lavori del Senato. È accaduto con gli emendamenti del relatore al decreto-legge sugli obblighi comunitari, riaccade ora con questi emendamenti, che saranno sicuramente in linea con quanto oggi previsto dal nostro Regolamento, non lo si potrà negare - privano gli stessi parlamentari del diritto di discutere, e vedersi anche bocciare, con i tempi dovuti, le proposte di modifica del testo in questione, ovviamente, nelle sedi deputate, ovvero nella Commissione difesa prima e nell'Aula subito dopo.

Fornire uno specifico quadro normativo di carattere anche sanzionatorio, a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e per evitare l'uso improprio da parte di terzi, istituendo una società per azioni a a totale partecipazione pubblica per gestire attività di carattere negoziale e gestionale, è sicuramente un compito di cui si può e si deve discutere. Non si può discutere però, di un testo introdotto in questo modo e che, seppur ha voluto esplicitamente escludere le attività della suddetta società nel campo immobiliare, non può soddisfare le esigenze di alcuno, se non dei nuovi nominati nel consiglio d'amministrazione della costituenda società. La creazione di una società *in house* del Ministero della difesa pone il problema di dover definire i rapporti con le strutture dello Stato già operanti nel settore, con riferimento sia a quelle interne allo stesso Dicastero, che a quelle relative a società pubbliche o a partecipazione pubblica. In particolare, per queste ultime, la necessità di evitare duplicazioni e conflitti di attribuzioni è maggiore che non nel caso delle strutture interne alla Difesa e presuppone un preventivo coordinamento delle attività. Nulla di tutto ciò è contenuto nei pochi commi introdotti dal voto della Commissione bilancio. Nulla più è scritto circa il coordinamento che le direzioni generali, nel disegno originario, potevano esplicare su detto organo, che oggi, nella formulazione che riceviamo, è semplicemente sottoposto al Ministro, senza sapere cosa ne sarà dei numerosi uffici che oggi si occupano delle stesse identiche cose. Nulla più è detto circa le sanzioni cui va incontro chi sfrutta in modo illegale gli stemmi e i loghi delle nostre Forze armate. È tutto sapientemente rinviato a un decreto del Ministro, che potrà o non potrà contenere queste disposizioni ma, come dicevo in precedenza, di certo conterrà i nomi dei membri del consiglio d'amministrazione, quindi poi dei sindaci, dei revisori, dei consulenti, e così e così via. Nulla è inoltre riportato circa le modalità con le quali il personale delle Forze armate, e non solo (anche i civili), potrà transitare in questa nuova società. È ipotizzabile - se non molto probabile - una corsa ad occupare posti nella nuova società da parte di militari, soprattutto alti ufficiali nella fase terminale della carriera, al fine di garantirsi un maggior numero di anni di servizio e indennità di trasferimento ad altro incarico. Al riguardo, avrei voluto proporre in Commissione difesa un'opportuna riformulazione dell'originario articolo, prevedendo magari modalità specifiche o requisiti minimi, al fine di consentire che possano passare in servizio presso la nuova società solo determinate figure in possesso appunto di requisiti specifici, acquisiti nel tempo e nelle more dello svolgimento del proprio lavoro, utili al raggiungimento dei fini che la costituenda società si prefigge. In particolare, sarebbe auspicabile escludere esplicitamente la possibilità che i vertici delle Forze armate che abbiano terminato o siano in procinto di terminare per intervenuti limiti di età, ai sensi della normativa vigente, la loro carriera, passino alla società in questione. Concludo, Presidente, palesando, a lei e a tutta l'Aula, la più profonda contrarietà del Gruppo Italia dei Valori sia verso il provvedimento in generale, iniquo e foriero solo di ulteriori disagi per i cittadini italiani, sia verso questo ennesimo colpo di mano che si sta operando a danno del settore della Difesa, che dal giorno dopo l'approvazione di questa finanziaria, con la scusa di snellire e semplificare procedure, avrà un altro carrozzone con compiti non chiari, almeno fino a quando il Governo non la smetterà di giocare a carte coperte,

Presidente, il bilancio e la finanziaria in esame dedicano uno spazio limitato ai temi della scuola e dell'università; diremmo uno spazio contabile senza alcuna prospettiva di tipo didattico e culturale. Sono semplicemente mantenuti i tagli di risorse triennali previsti dalla legge n. 133 del 2008, 8 miliardi per un triennio per la scuola, un miliardo e mezzo per l'università. Eppure, in convegni, conferenze stampe e interviste televisive, il Ministro e il Governo avevano rassicurato che i tagli per il 2010 sarebbero stati rivisti. Pertanto, la riforma delle superiori, che la 7a Commissione esaminerà la prossima settimana, ha come esclusiva premessa il completamento di quella che il ministro Tremonti definì la «sforbiciata», ovvero 130.000 posti in meno tra docenti e non. Il riconoscimento del merito per gli insegnanti migliori è rinviato al prossimo anno; il cosiddetto decreto salva precari, che l'Aula esaminerà nei prossimi giorni, di fatto, toglie ai precari i diritti previsti dal piano triennale di assunzioni della finanziaria 2007. La scorsa settimana il ministro Gelmini ha presentato con grande enfasi la riforma dell'università italiana; raccogliamo, come Gruppo del PD, l'invito ad un confronto serio nel merito, anche perché alcune delle proposte sono identiche a quelle indicate dal nostro disegno di legge sull'università, presentato ormai da parecchi mesi; ma con quali risorse la si finanzierà?

che all'avvio della discussione parlamentare, a garanzia della credibilità del processo riformatore che s'intende promuovere, corrisponda una disponibilità adeguata di risorse su un arco pluriennale, a cominciare da quelle che, entro poche settimane, dovranno essere garantite al fondo di finanziamento degli atenei per il 2010, senza le quali risulterà in molti casi impossibile la stessa predisposizione di bilanci di previsione in pareggio per il nuovo anno. Ci viene risposto dalla maggioranza che per il 2010 la riforma universitaria sarà finanziata con le risorse dello scudo fiscale; per il piano triennale, tuttavia, al di là della certezza delle entrate, quanti scudi fiscali prevede il Governo? Si dovrebbero poi aggiungere i 135 milioni tagliati alle scuole materne paritarie, che svolgono una funzione pubblica e unica nei piccoli Comuni, che si aggiungono ai 120 dell'anno scorso, non ancora distribuiti. Non era forse questo Governo - molto più di noi difensore della libertà educativa? Abbiamo dato a più riprese la disponibilità come Gruppo del Partito Democratico ad un patto di legislatura su scuola ed

ambiti troppo importanti su cui, durante la crisi, tanti Paesi come gli Stati Uniti e la Francia hanno previsto strategie ed investimenti importanti. La disponibilità è ancora intatta, ma non possiamo come opposizione diventare complici solo di un saccheggio di risorse. Sarebbe come rinunciare ad un messaggio di speranza e di futuro per i giovani di questo Paese.

nella finanziaria messa in campo per il 2008, venne fatta una normativa che penalizzava fortemente le aziende. Nello specifico, le penalizzava perché prevedeva la limitazione del 30 per cento della deducibilità degli oneri passivi che dovevano sostenere. Dovete sapere che queste aziende hanno una grossa immobilizzazione di capitali, perché con la stagionatura comprano a 60 giorni; giorni; pagando a 60 giorni tutto il materiale primario che poi devono tenere in stagionatura per un periodo che può arrivare anche oltre i 20 mesi, voi capite che hanno il capitale fermo.

prendiamoci tutti la responsabilità di fare un ragionamento giusto: le aziende in un momento come questo di crisi economica si vedono costrette ad andare

ho scoperto che se lavorassimo in maniera intelligente su questo emendamento - vi cito degli esempi - il comparto del prosciutto di Parma avrebbe un immediato beneficio di 25-30 milioni di euro. Delle 164 aziende, almeno la metà di queste, che hanno un indotto di 800 milioni di euro alla produzione, diventerebbero 1500. Sarebbe uguale per

Poi, quando è il momento di dare loro un aiuto concreto, non succede niente. Ho fatto una piccola ricerca storica: guardate che sono almeno 15 anni che il Governo ed il Parlamento non prendono atto e non si mobilitano per dare respiro a queste aziende. Ritengo che sia una cosa sbagliatissima. Sono mediamente piccole e medie aziende, non sono la classica Fiat: i salumifici sono entità che hanno mediamente 20, 30, 40 lavoratori.

particolare interna ai partiti, si suole dire che tutto va male e che tutto non funziona. Non è così! Va male quello che interessa dire che va male! E spesso e volentieri, quando si è

anche se il Presidente del Consiglio continua a ripetere che il peggio ormai è alle nostre spalle. Anche Dominique Strauss-Kahn, direttore generale del Fondo monetario internazionale, ha detto che la ripresa è ripartita prima del previsto, però ha aggiunto che c'è il rischio che sia senza posti di lavoro. Questo è uno dei tanti problemi che abbiamo di fronte e che questa finanziaria e questo bilancio non risolvono. In un contesto così problematico il bilancio del 2010 dovrebbe avere un valore politico aggiunto, invece parliamo continuamente di mancati finanziamenti; infatti, abbiamo visto che anche i rappresentanti della maggioranza hanno presentato circa il 20 per cento degli emendamenti (alcuni di questi sono stati annunciati anche questa mattina). Credo invece che con molta pacatezza e con molta ragionevolezza valga la pena di accogliere le parole che arrivano sia da parte sindacale sia da parte di Confindustria; entrambi questi mondi ci dicono che non c'è più tempo dobbiamo cercare di reagire. Vorrei porre l'attenzione su due aspetti: il mondo delle piccole e medie imprese e il mondo della famiglia, partendo proprio dalla famiglia. La spesa delle famiglie si è ridotta dello 0,5 per cento ed il reddito disponibile negli ultimi tre mesi si è ridotto dell'1 non solo, ciò che conta per lo Stato è che la famiglia italiana risulta la meno aiutata e incentivata in Europa. Infatti, mentre in Germania e Svezia si spende

Nonostante la crisi, la Francia e la Germania hanno registrato nel secondo trimestre 2009 una crescita del prodotto interno lordo dello 0,3 avendo puntato entrambe sul sostegno alla famiglia. Il quadro europeo ci dimostra che investire sulla famiglia vuol dire non solo guardare al futuro ma soprattutto sconfiggere la crisi. La famiglia è la forza della società. Stupisce molto che il Governo, che ha fatto della famiglia la sua bandiera, la paladina della campagna elettorale, parlando continuamente di quoziente familiare, adesso si sia dimenticato dell'esistenza della famiglia. Abbiamo presentato un pacchetto famiglia, abbiamo tentato di dare delle soluzioni. Siamo partiti dalla proposta del quoziente familiare ma abbiamo fatto anche proposte intermedie, che comportano minori risorse economiche e che potrebbero dare dare un sostegno, per esempio, alle famiglie che hanno al loro interno persone non autosufficienti o a quelle che hanno bisogno, avendo figli piccoli, di disporre di asili nido e di apposite comunità, così da consentire a entrambi i genitori, non solo al papà ma anche alla mamma, di lavorare, anche perché siamo il Paese che ha il più basso tasso di occupazione femminile. Di tutto questo, però, all'interno delle scelte dell'attuale Governo non c'è proprio nulla; è una sorta di silenzio assordante che fa paura, a fronte del quale le famiglie sono in un'attesa tranquilla, non rivoluzionaria, ma aspettano una scelta. Per quanto attiene invece il mondo dell'impresa, credo che anche su questo ci sia una sorta di confusione legalizzata. Il periodo natalizio è uno dei più propizi ai consumi. All'interno delle proposte di legge che abbiamo presentato ce ne é una per la riduzione e l'abbattimento dell'imposizione sulla cosiddetta tredicesima mensilità.

terrebbe insieme politica familiare e politica economica, però di questo non sembra ci sia traccia né all'interno della finanziaria né tantomeno nelle intenzioni di questo Governo. Voglio citare una scelta fatta in Francia e sulla quale nella terra dalla quale provengo (la Brianza) si sta discutendo proprio perché viene ritenuta proficua. In Francia è stata soppressa la *taxe* *professionnelle*, che è l'equivalente della nostra IRAP. Le piccole aziende, che hanno assunto 500.000 nuovi lavoratori, non hanno così pagato i contributi; questo ha rappresentato un volano per l'economia. In Italia cosa si sta facendo? Attualmente sono circa un milione i lavoratori coinvolti dalla cassa integrazione e le imprese che nel corso di tutto il 2009 si stima faranno ricorso agli ammortizzatori in deroga sono circa 36.000. I decreti di cassa integrazione straordinaria da gennaio ad agosto 2009 riguardano 1.779 aziende e 2.552 siti produttivi. Confindustria sostiene che ci sia un rischio di chiusura per un milione di aziende. Si tratta di dati allarmanti, che vanno detti con un tono di voce basso, perché riguardano persone che perdono il posto di lavoro e che non hanno più speranza per il lavoro futuro. Occorrerebbero delle misure in grado di dare liquidità momentanea per il periodo di crisi: un atto di fiducia verso l'industria italiana che non è presente però in Per questo abbiamo presentato un disegno di legge e un emendamento sull'estensione del regime dell'IVA per cassa per consentire alle piccole e medie imprese di versare l'IVA allo Stato solo al momento dell'incasso. Ritengo, inoltre, necessario e urgente aiutare i giovani con meno di 35 anni che vogliono avviare un'impresa e anche per questo abbiamo presentato un emendamento. Proponiamo Proponiamo di pagare un'imposta del 12,5 per cento per i primi tre anni di attività; è la stessa imposta che paga chi vive di rendita finanziaria e, quindi, crediamo che sia il minimo che lo Stato possa consentire.

oggi, per consentire al nostro Paese di crescere domani. Usando le parole della poetessa Alda Merini, a cui va il nostro commosso saluto,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, sento innanzitutto il piacere e il dovere di sottolineare che condivido l'impostazione che il Governo dà a questa finanziaria,

di suggerire e di fare delle considerazioni che non sono in distonia con l'impostazione del Governo, ma che vanno nella direzione di dare suggerimenti per migliorare da assumere per il Mezzogiorno d'Italia. Da uomo del Mezzogiorno d'Italia, vorrei soffermarmi su questo aspetto e sottolineare alcune considerazioni che ci riportano all'analisi della fase storica particolarmente difficile, in cui risultano amplificate le grandi sofferenze che attualmente investono per la verità tutto il Paese, ma soprattutto il Mezzogiorno, proprio in ragione del suo storico ritardo nello sviluppo. La scuola, la giustizia, la sicurezza e la pubblica amministrazione funzionano infatti nel Sud del Paese assai peggio che nella media nazionale. In altri termini*,* se si può ben affermare che il ritardo nello sviluppo del Mezzogiorno sia uno dei problemi più gravi d'Italia, corrisponde altresì al vero che il ritardo in parte è dovuto proprio al fatto che non sono state adeguate in quantità e soprattutto in qualità le politiche sino ad oggi attivate

Per più di un decennio, i Governi hanno dunque fissato un obiettivo di spesa in conto capitale nel Mezzogiorno condiviso fra tutte le forze politiche e confermato per ben tre legislature, anche se ridotto nell'ultima, che poi alla prova dei fatti è risultato disatteso. Gli obiettivi di spesa nel Sud non sono mai stati realizzati e la spesa in conto capitale è infatti aumentata nel Centro Nord, non nel Mezzogiorno: lo attestano i dati registrati dal 2001 al 2006, dai quali emerge che la spesa del Mezzogiorno è passata da 21 a 22,2 miliardi di euro

Di fronte a queste evidenze, occorre ribadire ancora una volta che la questione del Mezzogiorno è questione nazionale, non regionale, anzi, è primaria per il nostro Paese. Non possiamo accettare che il Paese si divida per una crescente dualità, poiché a conti fatti esso è senza dubbio in debito

Se non è pienamente condivisibile quanto detto dal Ministro dell'economia in una recente occasione, relativamente al fatto che l'unificazione d'Italia, compiuta con le baionette dell'esercito sabaudo, non sarebbe stata un'operazione totalmente positiva, è pur vero che i 150 anni di unità nazionale non hanno risolto il ritardo di sviluppo né hanno alterato le profonde ragioni del disagio sociale. Tuttavia, per affrontare con onestà intellettuale il dibattito sui temi del Mezzogiorno alla luce della crisi economica in atto, occorre partire da un'imprescindibile premessa di merito: gran parte dei problemi economici dell'Italia,

Il Nord, infatti, anche in questa crisi riesce comunque a difendere la coesione ed il tessuto produttivo, mostrando una sostanziale tenuta del sistema sociale con un fortissimo aggravio del bilancio dello Stato; in molti settori il Nord ha persino problemi di limiti di crescita, in particolare per mancanza di manodopera qualificata. Di converso, il Sud rischia di sprofondare ancor più e di essere ulteriormente marginalizzato dalla crisi in atto, in un contesto di crescenti difficoltà indotte dalle globalizzazione. Le cifre del Sud, come primo problema nazionale, sono evidenti a tutti, anche se qualcuno finge di non vederle, e mi riferisco - com'è ovvio - al PIL per abitante, alla disoccupazione, al deficit infrastrutturale.

e di occupazione, non cresce nemmeno l'Italia; e l'egoismo, per la verità, non paga. Sul punto, perciò, occorre ribadire ancora una volta che non è per nulla condivisibile la tesi per cui le risorse destinate al Sud sono sprecate, in quanto non ci sarebbero le energie positive e le capacità di utilizzarle al meglio; una tesi che una certa opinione opinione distorta tende sempre più ad accreditare, sull'onda dei tanti esempi pur presenti - con onestà intellettuale dobbiamo riconoscerlo - di malaffare, di sprechi, se non di vere e proprie ruberie. La nostra opinione è infatti che il Sud abbia in sé, in particolare nelle nuove generazioni, le energie positive per ripartire, fatto che è dimostrato dai tanti esempi di distretti industriali e di singole eccellenze di nicchia, per le quali occorre fare ogni sforzo per assicurare loro un tranquillo sentiero di crescita e di sviluppo. Basti pensare al settore del turismo. Tante città del Sud sono diventate una destinazione turistica sofisticata; non solo, alcuni dei migliori prodotti agricoli di qualità vengono dal Sud. In Puglia, soprattutto, che segna da anni un buon tasso di crescita; non altrettanto, per la verità, fanno la mia Campania e la Calabria. Tutto questo ci dimostra che non esiste un solo Sud, ma diverse realtà locali, dove non mancano i germogli di un percorso di sviluppo civile ed economico. Dall'inizio della legislatura, impegnato su problemi ovviamente importanti, ma - mi sia permesso - più contingenti rispetto al tema del divario Nord Sud (come la crisi finanziaria, il terremoto dell'Abruzzo, il G8), il Governo non ha potuto dedicare la necessaria attenzione allo sviluppo del Mezzogiorno, che è il problema dei problemi, perché da esso dipendono molti altri, a partire dalla criminalità organizzata. In tal senso, sebbene le decisioni prese nello scorso luglio abbiano rappresentato l'inizio di una svolta positiva della politica per il Sud, occorre ora tradurre tali strategie in atti più concreti, progetti attuativi e precise responsabilità. Per la verità, dei primi 4 miliardi e 300 milioni di euro che sono stati assegnati alla Sicilia da parte del CIPE a fine luglio, il 43 per cento sarà destinato ad opere strategiche. Sono stati evitati finalmente i finanziamenti a pioggia ed è stata data priorità ai finanziamenti in conto capitale, per recuperare i ritardi infrastrutturali. Questa - io credo - è la strada giusta, ma occorre vigilare perché sia effettivamente così. Gli annunci e la riunione del CIPE di fine luglio scorso sono stati in questo senso un fatto storico. Vi è stato l'avvio della discussione del nuovo piano decennale per il Sud, con la previsione anche della Banca del Mezzogiorno (la Banca del Sud), che è di antica memoria e che finalmente abbiamo visto avviarsi alla sua realizzazione, nonché del nuovo ente di coordinamento degli investimenti e delle azioni di sviluppo a favore del Mezzogiorno. Si tratta di segnali certamente non negativi, ma che si ha necessità di incrementare e di avviare, per far sì che la spesa nefanda che hanno fatto le amministrazioni regionali di sinistra (a cominciare dalla Campania) possa finalmente essere orientata verso lo sviluppo del Paese e verso un'azione armonica e concreta rispetto all'obiettivo

sull'opportunità del federalismo fiscale, che recupererà la responsabilità degli amministratori. Voglio dirlo al vice ministro Vegas e al Governo: attenzione all'ipotesi di riduzione dell'IRAP. Noi siamo perfettamente d'accordo e siamo perfettamente orientati in quella direzione. Ma attenzione: l'IRAP deve essere ridotta

Com'è possibile immaginare lo sviluppo del Mezzogiorno, delle imprese del Mezzogiorno, se non lo aiutiamo a ridurre questa imposta nefanda e improduttiva? Nella riduzione dell'IRAP bisognerà bisognerà tener conto di queste esigenze e di queste realtà del territorio; la riduzione dovrà pertanto essere differenziata tra le imprese del Nord e le imprese del Sud, per recuperare questo gap. Altrimenti, avremo ancora di più l'affossamento dell'economia e l'affossamento dell'aspirazione del popolo del Mezzogiorno,

la valutazione che ho già espresso. Nel corso del suo intervento, il senatore Torri ha usato un paio di espressioni che non sono semplicemente al limite, ma sono da evitare nei lavori parlamentari e nel dibattito in quest'Aula.

*(PD)*. Signor Presidente, non svolgerò tutte le considerazioni che riguardano gli effetti della manovra finanziaria sulla politica estera e richiamo a tal fine la relazione di minoranza che abbiamo presentato in Commissione. Mi soffermo nel mio intervento esclusivamente su due punti nonché su alcune considerazioni e domande che voglio lanciare in primo luogo al vice ministro Vegas e al Governo,

C'è un dato che di per sé è molto evidente: si passa dagli 848 milioni di euro della finanziaria del

il 16 novembre prossimo il Presidente del Consiglio, piuttosto che presentarsi al tribunale di Milano, dovrà andare alla Conferenza internazionale sull'alimentazione per spiegare e giustificare il motivo per cui la parola data dall'Italia non conta nulla; naturalmente, ciò richiederà una presenza ed un impegno del tutto particolari. Aggiungo che di nuovo siamo in presenza di una posizione del Governo che rifiuta di considerare il contributo italiano alla lotta contro le pandemie, cioè alla lotta contro la malaria,

di un impegno strutturale e permanente del nostro Paese, se vogliamo partecipare e appartenere, avendo qualche diritto di parola e una voce ascoltata, alla comunità internazionale.

vice ministro Vegas, lei sa che per la prima volta da molti anni questa finanziaria non rifinanzia i fondi per le missioni internazionali. Fino al 2003, le missioni internazionali erano finanziate attraverso il Fondo per le spese impreviste. Da allora, le missioni sono entrate di volta in volta nelle leggi finanziarie fino a quando, nel 2007, è iniziata una programmazione triennale con l'istituzione di un Fondo, finanziato con circa un miliardo di euro all'anno e poi integrato di volta in volta, che ha coperto il triennio 2007-2009.

indicherà di volta in volta? È su questa base che decideremo se restare o no in Libano? Se restare o non restare (e come restare) nelle altre missioni internazionali nelle quali siamo impegnati? È un punto molto importante e molto delicato

che consideri come un fatto permanente, e non come una spesa imprevista, il far fronte ai propri impegni internazionali, il partecipare nella comunità internazionale agli obblighi che ci assumiamo e a contribuire in base e in ragione delle nostre forze e delle nostre possibilità a uno sforzo collettivo della comunità internazionale per la pace e la sicurezza.

un passo indietro significativo rispetto a un'idea politica del nostro Paese, del suo futuro e della sua collocazione nel mondo. Concludo, signor Presidente, ribadendo che, quando parlo di tali argomenti, non posso non pensare alla politica, cioè al fatto che, se vogliamo affrontare questi problemi, abbiamo bisogno di trovare uno spazio. Questi problemi, infatti, non si possono affrontare sulla base dei sondaggi di opinione o di un'impostazione populistica. O noi troviamo uno spazio dove riuscire a prendere una distanza dalla cronaca e dagli umori mediati e ad assumerci le responsabilità su un terreno che, naturalmente, non è quello sul quale si ricevono gli applausi di questa o quella categoria; oppure, noi comprometteremo seriamente

o su come sia assolutamente condiviso dalla Lega Nord l'obiettivo primario di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica. A tal proposito, mi permetto di consigliare caldamente, a chi non avesse avuto modo di seguirlo in diretta, di leggere l'intervento pronunciato ieri sera in Aula dal collega Massimo Garavaglia, che ritengo estremamente educativo non solo per chi come noi svolge il proprio compito nelle Aule parlamentari. La Lega Nord nell'affrontare il lavoro propedeutico alla definizione degli obiettivi che rappresentano il nostro contributo a questa manovra finanziaria ha focalizzato l'attenzione su alcuni temi che ritiene assolutamente prioritari.

e dell'Aula quanto la Lega Nord propone attraverso un emendamento che vuol essere un importante contributo alla richiesta di sicurezza nel trasporto delle merci pericolose. Si è parlato molte volte in quest'Aula di questo argomento a seguito della tragedia di Viareggio. Riconosciamo sicuramente le buone intenzioni e gli impegni già espressi dal Governo e ribaditi anche recentemente dal Ministro delle infrastrutture.

Ricordiamo allora alcuni numeri sul GPL. L'Italia settentrionale ha consumato dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009 circa 1.200.000 tonnellate di GPL propano,

Questo rappresenta un pericolo assolutamente costante, che potrebbe essere evitato ricorrendo ad una via alternativa che è quella che proponiamo oggi all'attenzione del Governo e dell'Aula: quella del trasporto fluviale, utilizzando una flotta di chiatte gasiere per il trasporto di GPL dal mare al centro della Pianura padana. Pensiamo che una di queste gasiere toglierebbe dalla strada 90 autobotti. Dal centro della Pianura padana poi il GPL può essere sicuramente trasferito nei centri di consumo con una percorrenza media inferiore ai 200 km (come richiesto, peraltro, in Europa dalla normativa tedesca). Il trasporto stradale del GPL è in assoluto il più pericoloso: transita all'interno dei centri abitati; spesso, purtroppo, non vengono rispettati i tempi di sosta e di guida degli autisti; viaggia con percorrenze medie di oltre 1.000 chilometri.

ma l'incidente di Viareggio ha messo in evidenza come anche tale sistema di trasporto, pur prevedendo maggiori garanzie di sicurezza, ha sempre degli elevati tassa di pericolosità. di pericolosità. Pertanto, riteniamo che il trasporto fluviale di GPL debba assolutamente disporre di incentivi, come avviene in tutti i Paesi europei, dove viene premiata l'eliminazione dei pericoli derivanti dal trasporto.

al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, ma si potrebbe anche pensare, con un impatto veramente minimo, a un aumento di 4 euro per tonnellata dell'accisa gravante sul GPL ad uso per combustione ed autotrazione.

la finanziaria *light*, leggera, quasi evanescente approvata dal Consiglio dei ministri, non affronta nessuno dei gravissimi problemi del Paese reale, che restano fuori dalle finzioni e da una mistificazione mediatica, ordinata dai soliti lorsignori che controllano, direttamente o indirettamente, i mezzi di informazione, soprattutto le televisioni. Costoro tendono a bollare come nemici dell'Italia tutti coloro che non vedono come imminente l'uscita dal tunnel della crisi. Non sono disfattiste ed anti-italiane le famiglie che continuano a faticare ed a ricorrere a grandi sacrifici per mandare i figli a scuola, oppure coloro che sono costretti a contrarre sempre più debiti ricorrendo al credito al consumo ed alle carte *revolving*, vere e proprie trappole piene di interessi Non sono disfattisti quegli imprenditori che da mesi invitano il Governo a studiare misure anticicliche ed esortano a mettere soldi veri per l'*exit strategy*, non quei soldi finti che si spostano come i cannoni del Ventennio da un avamposto all'altro.

Per rilanciare l'economia non basta pensare alle imprese con il taglio, pur lieve, dell'IRAP. Con la difficoltà ad esportare a causa dell'euro forte, occorre rilanciare la domanda interna ed offrire più redditi alle famiglie, sempre più tartassate da una pressione fiscale aumentata dal 42,8 al 43 Gli ultimi dati di Findomestic sui consumi e la fiducia degli italiani, che ad ottobre torna a calare facendo diminuire le previsioni di risparmio, non fanno altro che confermare ed aggravare le prospettive sulla pesante contrazione dei consumi

L'andamento dei consumi incide anche sulle spese anelastiche, come gli alimentari, e la ripresa del PIL dello 0,7 per cento prospettata per il 2010 risulta marginale. L'onda lunga di cassa integrazione e disoccupazione dovrà ancora dispiegare i suoi effetti, contribuendo così ad abbattere ulteriormente il potere d'acquisto delle famiglie, già ridotto ai minimi termini. Il Governo, piuttosto che pensare a come sgravare gli oneri fiscali alle imprese, dovrebbe varare con urgenza un intervento teso ad incrementare il potere d'acquisto delle famiglie, con una detassazione del reddito fisso per almeno 1.200-1.500 euro annui, detassare le tredicesime offrendo misure di sostegno per il reddito dei precari ed un calmiere sui prezzi. Le banche, responsabili della crisi per la sfrenata avidità, non aiutano il Paese a trovare vie di uscita con una restrizione del credito, confermata perfino dal Governatore della Banca d'Italia in occasione della Giornata del risparmio, che qualcuno ha ribattezzato Giornata del debito. I dati ieri dalla Banca d'Italia segnalano che un terzo delle aziende ha avuto un inasprimento delle condizioni di finanziamento. Il 61 per cento cita tra i motivi di tale peggioramento un maggiore costo o una richiesta di garanzie più elevate; il 28,2 per cento il non accoglimento delle proprie domande di nuovi finanziamenti; il 22,1 per cento una richiesta di rientro, anche parziale, dei fidi in essere. Queste ultime due modalità sono indicate con maggiore frequenza dalle aziende con meno di duecento dipendenti. Questo sistema bancario, che ha contribuito a generare la crisi e che eroga crediti allegri con criteri amicali ai sodali come Zunino di Risanamento, continua a negarlo quindi alle piccole e medie imprese che hanno bisogno di piccoli fidi di 50.000-100.000 euro per continuare l'attività e non licenziare 15-20 dipendenti. quegli stessi banchieri che, abrogato il pizzo della commissione di massimo scoperto, gli hanno solo cambiato denominazione, continuando a praticare l'usura legalizzata a danno delle piccole e medie imprese e delle famiglie. I recenti interventi legislativi in materia di costo degli affidamenti degli scoperti hanno solo in parte conseguito gli effetti sperati. Le banche hanno cambiato la struttura delle commissioni, anche per recuperare componenti di reddito non più applicabili per legge. Non lo dice il senatore Lannutti o un'associazione, bensì il governatore della Banca d'Italia Draghi. La questione creditizia e la gestione del credito e del risparmio diventano così questioni di emergenza nazionale, con banchieri che continuano indisturbati a fare il comodo proprio e a dare ordini agli esecutivi di qualsivoglia colore politico, non pagando mai il conto; anzi facendo peggio di prima, come risulta dall'esposizione

di una politica economica profondamente sbagliata. È il grande capolavoro del Governo, che è riuscito ad aumentare il debito pubblico italiano che nell'ottobre scorso gravava per 79.500 euro sulle spalle di ogni famiglia e lo ha aumentato di ben 4.178 euro in soli 10 mesi. Questa enorme massa di debito pubblico si poteva ridurre, sia utilizzando le dismissioni di oro e riserve della Banca d'Italia, come hanno fatto tutti gli altri Paesi dell'area euro, sia attuando politiche economiche di dismissioni dell'enorme patrimonio del demanio, neppure ben censito, o riducendo la spesa pubblica, che continua a dilatarsi per finanziare enti inutili, le consuete clientele, mentre il salvataggio di Alitalia il cui costo, pari a 3 miliardi di euro, a favore di capitani coraggiosi, è stato addossato alla fiscalità generale.

nel 2010 e al 117,8 per cento nel 2011. Gli oneri del debito sono pari al 5 per cento del prodotto interno lordo: un livello superiore a qualsiasi altro Paese. A causa di questo fardello, l'Italia «non può finanziare investimenti in formazione e in infrastrutture di cui avrebbe bisogno». Il PIL scenderà quest'anno del 4,7 per cento, rendendo ancora meno sostenibile il rapporto con il debito, e solo nel 2010 dovrebbe far registrare un timido più 0,7 per cento, nel 2011. L'unica ricetta possibile per l'Italia è di tornare ad un elevato avanzo primario «in modo da riportare nuovamente il debito su una china discendente». Preoccupazioni analoghe sono state espresse anche dal rapporto del Fondo monetario internazionale, che punta il dito sullo stretto rapporto esistente tra l'alto debito e le basse potenzialità di crescita. L'Italia, insomma, sarebbe in piena sindrome giapponese e per uscirne, secondo il Fondo monetario, dovrebbe mettere in atto una manovra pari al 4,8 per cento del PIL per risollevare l'avanzo primario del Paese. Quando il Governo, però, per assecondare i *desiderata* di banche, assicurazioni, monopoli e cartelli, svuota e rinvia uno strumento di civiltà giuridica, un contrappeso alla protervia dei potentati economici come la *class action*, sostituita - lo dico per l'ennesima volta - con la «*farce action*», una farsa del ministro Brunetta, una vera e propria presa in giro, che meriterebbe di essere portata in giudizio come abuso della credulità popolare, ed avvia tutta una serie di controriforme in alcuni settori, faticosamente liberalizzati dal ministro Bersani, offrendo la sua ala protettrice ad alcuni ordini e professioni messe sotto la lente dell'Antitrust, non aiuta il Paese ad uscire dalla crisi. Quando il Governo continua ad ignorare i bisogni di tanti creditori, spesso piccole e medie imprese che vantano crediti per 40 miliardi di euro nei confronti della pubblica amministrazione, evitando di studiare e concordare strategie, anche con la Commissione europea, per trovare soluzioni, è affetto da una miopia economica oltre che politica. In un'epoca dove le banche, tornate a scommettere con i derivati,

di anticipare le somme vantate nei confronti della pubblica amministrazione? Sono domande lecite che rivolgiamo da tempo invano al Ministro dell'economia e alla maggioranza e veniamo accusati di lesa maestà. Crediamo che si possano studiare strategie condivise per far uscire il Paese dalla grave crisi economica ed abbiamo avanzato molte proposte, riassunte anche dal presidente Baldassarri nella controfinanziaria, che mi risulta sia stata bocciata dalla sua stessa maggioranza, come l'utilizzo poco trasparente di oltre 35 miliardi di euro a fondo perduto. Per queste ragioni, signor Presidente, esprimiamo un giudizio molto severo su una finanziaria sbagliata,

*(PdL)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatrici e senatori, la discussione e il varo della finanziaria 2010 avvengono nell'ambito di uno scenario internazionale che appare meno cupo e difficile di quello che aveva contraddistinto, nello scorso mese di luglio, l'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria e la manovra attuata con il decreto-legge 1° Il complesso dei provvedimenti di politica finanziaria, compresa anche la Nota di aggiornamento del DPEF, discussa dal Parlamento un mese fa, si colloca in un momento di incertezza, che non riguarda però l'andamento della crisi bensì l'evoluzione della ripresa. Appare infatti ormai acclarato il fatto, confermato da molteplici elementi e segnalato dagli istituti di ricerca, che la ripresa in atto appare più consistente di quanto si potesse prevedere. Negli Stati Uniti la crescita del prodotto interno lordo è stata del 3,5 per cento nel terzo trimestre e lascia intravedere uno slancio dell'economia tale da indurre già a un risultato positivo del PIL nel 2010, oltre che a contenere, a livelli inferiori rispetto alle previsioni, il calo del medesimo parametro nell'anno in corso. Se si pensa che nel trimestre precedente il prodotto lordo è stato ancora negativo dello 0,7 per cento, si può misurare la rapidità con cui quella che resta la più grande economia mondiale ha ripreso slancio; la più grande economia mondiale, cui noi siamo legati nel *trend* anche nella nella nostra qualità di secondo Paese esportatore d'Europa. È inevitabile che tale vigore si ripercuota, pur con tempi e modalità differenti, sull'intero sistema economico mondiale e, dunque, su quello italiano, che già presenta segnali di inversione nella fiducia dei consumatori, negli indicatori che anticipano gli ordini e la produzione industriale, persino nella seppur lieve ripresa dell'indice dei prezzi - inequivocabile segno della ripresa dei consumi tornato in positivo dopo un decremento nei mesi di giugno e luglio. Restano le difficoltà legate al livello occupazionale, anche se il ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali - garantiti con tempestività dal Governo - ha permesso di attenuare la caduta di attenuare la caduta dell'occupazione e l'aumento del bacino dei disoccupati. Non è stato così per molti altri Paesi, segnatamente vorrei ricordare Spagna e Regno Unito, in cui la crisi occupazionale ha indotto un calo dei consumi indotto un calo dei consumi interni e dell'intera economia, facendo avvitare quei Paesi in una spirale recessiva molto più pesante della nostra. Siamo fortunatamente immuni dalle esaltazioni del nazionalismo economico che, nell'Europa unita, apparirebbero certamente risibili, e tuttavia è curioso curioso rimarcare l'enfasi con cui i media inglesi hanno sottolineato il fatto che il Regno Unito sia stato colpito da un calo su base annua del 5,2 per cento del PIL, con una serie negativa che dura ormai da sei trimestri, determinando un sorpasso dell'Italia come non avveniva da più di 15 anni. Da parte di molti media italiani si è preferito signorilmente sorvolare su questa notizia, forse per non essere costretti ad evidenziare quello che è indubbiamente un successo di tenuta del nostro Paese, ma anche delle politiche anticrisi messe in atto a più livelli dal Governo. Con la legge finanziaria e con il bilancio 2010 come bene esplicato dalle relazioni dei relatori Latronico e Saia che ringrazio - e con il quadro previsionale pluriennale che ne discende, si delinea la condizione dei conti pubblici in una prospettiva di ripresa. La scelta del Governo di impostare un provvedimento snello ma esaustivo è indubbiamente legata anche alle difficoltà di avventurarsi in previsioni circostanziate sull'andamento della congiuntura. Sulla basi degli elementi disponibili non si possono fare previsioni affidabili circa il ritmo della crescita. Il termine è ancora prudenza. Vorrei ricordare che si parla di una crisi non a forma di V, ma - vi è questo rischio - a forma di nel senso che la ripresa attuale potrebbe ricreare una grande bolla a seguito della liquidità immessa sul sistema finanziario e quindi sulle grandi banche; il rischio che questa liquidità rigeneri una bolla finanziaria, e quindi un nuovo crollo, è ancora oggi paventato da molti indicatori. Quindi, vi è la necessità di di un percorso di risanamento che sia condiviso da tutti gli Esecutivi a livello europeo e

La domanda sottesa, rispetto alle scelte da fare nel momento in cui gli elementi essenziali per una previsione fondata saranno reperibili, è quali siano le riforme necessarie a sostenere il sistema economico e produttivo. Naturalmente su questo resta automaticamente da definire l'aspetto della riduzione della pressione fiscale, elemento di programma

Tutto ciò non può prescindere - ad esempio - dall'attuazione di un corretto federalismo amministrativo e fiscale che giunga a responsabilizzare i diversi livelli di governo rispetto alle entrate e alle spese, così come previsto dalla Costituzione, evitando che vi sia una distorsione legata al ruolo di ultima istanza che le casse statali svolgono nei confronti degli enti locali in difficoltà di bilancio. Ed in tale quadro occorrerà, in un'ottica di lungo periodo, ripensare una politica fiscale che non sia unicamente orientata ad acquisire le risorse pubbliche, ma che sia strettamente collegata ed armonizzata con le politiche pubbliche, nella consapevolezza che ogni prelievo risulta distorsivo del mercato e va dunque valutato in ragione del suo impatto. Si tratta anche di modernizzare il Paese, di prendere atto del superamento di alcuni modelli che sono stati la caratteristica degli anni '70. Mi riferisco alla politica dei redditi basata sulla progressività delle aliquote, aspetto ormai completamente superato perché le moderne tecnologie, la mobilità delle persone fanno sì che solo una fascia di mezzo rientri nel sistema di applicazione delle imposte dirette sulla progressività delle aliquote. Quindi, vi è la necessità di spostarsi su un sistema di imposte in cui la tassazione sia essenzialmente sui consumi. Solo in questo modo si può anche unificare e riequilibrare il nostro sistema fiscale ed essere anche meno velleitari nel sistema di tassazione, diminuendo l'evasione che è ancora alta nel nostro Paese. La scommessa è che, grazie anche alla riforma *in itinere* delle norme di la contabilità pubblica ed alla ancor più rilevante riforma del federalismo, si riesca a creare un sistema fiscale, atto a sostenere la ripresa economica. Nell'ambito di un ripensamento generale delle politiche fiscali si dovrà anche valutare l'opportunità di intervenire con misure specifiche sui settori trainanti della nostra economia, che erano considerati settori maturi; ma la forza del nostro Paese -avendo già detto prima che è il secondo Paese esportatore d'Europa

L'Italia è l'ultimo Paese dell'Europa occidentale ad aver conservato una forte specificità nel settore manifatturiero tessile-abbigliamento in particolare, che conta oltre un milione di occupati su tutta la filiera. In considerazione degli evidenti segnali di ripresa che si colgono a livello internazionale, occorre prevedere un sostegno volto a rafforzare la competitività di tutto tutto ciò che fa sistema di filiera. Sono questi i temi che dovranno essere discussi in un confronto sereno tra Governo e Parlamento, ma nello stesso ambito della maggioranza, per aiutare

colleghi, caro senatore Saia**,** non so se le risorse richieste per la sanità sono troppe, come lei giustamente ha detto e la ringrazio perché almeno ha citato il tema. Sicuramente non se ne vedono in questa finanziaria. Sicuramente nelle tabelle di questo bilancio si vedono solo dei tagli, ma non si vedono risorse aggiuntive per la sanità. Tagli che suggeriscono l'idea che comunque si mette in discussione il ruolo sociale della sanità stessa in Italia; ruolo che sappiamo importante per garantire non solo l'accesso universalistico e solidaristico, ma anche perché è un modo di redistribuzione del reddito: tutti si possono curare nello stesso modo. Questo è il principio sancito dalla Costituzione, invidiato da tutto il mondo ed interpretato dal nostro sistema sanitario nazionale. Continui tagli trasversali della sanità mettono in discussione questo modello, ancor di più se consideriamo le parole del ministro Sacconi nel Libro bianco, che parla di universalismo selettivo. Quando l'universalismo è selettivo significa che qualcuno da quest'universalismo rimane fuori. Non vorremmo che a rimanere fuori fossero sempre i soliti, cioè quelli che alla fine hanno meno possibilità di accedere ai servizi efficienti e di maggior qualità.

siamo appunto trovati in Commissione sanità a parlare di legge finanziaria senza disporre di nessun elemento di riferimento nella legge; parallelamente Regioni e Stato stavano discutendo del Patto sulla salute. Anzi, a dire il vero avevano interrotto la loro discussione, un fatto gravissimo perché sappiamo bene che per mantenere questo meccanismo di efficienza del sistema sanitario ed anche di responsabilità delle Regioni, il rapporto tra Stato e Regioni è fondamentale proprio perché il nostro è un sistema di federalismo sanitario. L'aver interrotto in modo unilaterale da parte del Governo tale rapporto è stato un atto gravissimo. Mentre discutevamo in Commissione si consumava parallelamente questo atto che, per fortuna, è stato recuperato in data 23 ottobre attraverso la sigla di un patto, che prevede alcune cifre ed alcuni orientamenti, di cui però non c'è nessuna traccia in questa finanziaria. allora contenti che lo Stato abbia recuperato finalmente in modo saggio un rapporto con le Regioni, senza le quali non si fa la sanità in questo Paese. Siamo anche contenti che si siano previste le risorse aggiuntive che le Regioni chiedevano: circa

non sappiamo però come la promessa della copertura di queste spese verrà mantenuta; non so se vi sarà qualche emendamento ulteriore del Governo, ma al momento non c'è traccia di come questa promessa, questa sigla fra Regioni e Stato, verrà onorata dal Governo. per il 2010 possa essere coperta dalla solita *una tantum,* dallo scudo fiscale, non sappiamo poi come verranno onorati i patti fatti con le Regioni per il 2011 e 2012. Penso che in merito a tale aspetto, anche se stiamo facendo un po' di retorica, una risposta ci debba essere data

però questo patto per la salute che è stato siglato, ad oggi, in piena discussione finanziaria, quindi non ancora coperto, non prevede nemmeno gli obiettivi che le Regioni dovranno porsi.

non possiamo prevedere sempre più risorse rincorrendo le spese delle Regioni, questo è ovvio; dobbiamo quindi spingere le Regioni ad un maggiore risparmio, a recuperare le spese inutili, ad una maggiore efficienza. Abbiamo discusso tanto di come realizzare tale obiettivo, ma in questa finanziaria non c'è traccia di nulla, non ce ne è traccia neanche negli altri provvedimenti del Governo, dove di sanità se ne parla sempre in modo sporadico, in provvedimenti spesso*omnibus* di cui si fa fatica a rintracciare la logica. Noi vogliamo avanzare perché nella sanità vi sono grandi problemi e uno di questi, uno degli ambiti dove si annida la maggiore spesa inutile, è l'inappropriatezza delle prestazioni. Non c'è solo la corruzione

Se riuscissimo a ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni, per esempio modificando, come suggeriamo da tempo, il sistema del rimborso DRG penso faremmo qualcosa di assolutamente utile. Non basta più il rimborso quantitativo, bisogna parametrare la qualità con cui le prestazioni vengono effettuate nei nostri ospedali. Quindi, il rimborso deve tenere conto anche dell'efficienza, della qualità, dell'accoglienza, delle liste di attesa che le nostre strutture sanitarie offrono. dare a tutti lo stesso rimborso, bisogna integrarlo: altrimenti il sistema DRG incentiva l'inappropriatezza della spesa, le prestazioni per fare *budget*, fino ad arrivare a storture come quelle che abbiamo visto, a veri e propri atti illegittimi, anche di delinquenza, contro lo Stato. È chiaro che questo discorso di inappropriatezza si accompagna un necessario controllo della spesa sanitaria, ma non c'è niente su questo. Ci mettiamo nuovi soldi e sono contento perché le Regioni lo chiedono, perché serve per riadeguare il Nord e il Sud. Sappiamo che la sanità va a un regime diverso e, quindi, bisogna riadeguarla perché il sistema non può essere diverso al Nord e al Sud: i nostri cittadini cittadini sono uguali in Calabria come in Lombardia e bisogna smetterla con il fenomeno del turismo sanitario. Questo si ottiene anche con un controllo della spesa, e non possiamo sempre invocare il federalismo fiscale come momento di approdo e di risoluzione di tutti i problemi: cominciamo a farlo prima. a farlo prima. È inutile tagliare i livelli di assistenza essenziali, lo trovo assolutamente negativo. Noi dobbiamo invece mantenere dei buoni livelli di assistenza per i nostri cittadini proprio per evitare che ci siano quelli di seria A e quelli di serie B, ma dobbiamo anche inserire il tema del controllo del costo delle prestazioni da parte delle Regioni, cosa che non è stato fatto in passato, ma che, noto, non viene fatto neanche ora. In conclusione, abbiamo il problema delle risorse che, ripeto, non so come verranno coperte, ma anche il problema degli obiettivi, che non sono chiari.

A. Penso che la finanziaria sia assolutamente inadatta ad affrontare la situazione sociale, che vede le nostre famiglie esposte a una crisi molto pesante. Spero che alla fine i soldi di i soldi di coloro che hanno evaso il fisco rientrando nel nostro Paese diano una mano a chi le tasse le ha sempre pagate e continua a farlo, anche se oggi non ha più i soldi per pagare l'affitto e, magari, non ha neanche più la casa. Spero in un atto di

Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, chiedo un attimo di attenzione su due proposte che andremo a valutare, riguardo il finanziamento del sistema universitario. Una riguarda l'IVA che gli atenei sborsano per l'acquisto di materiale amministrativo e didattico, funzionale alle attività primarie e di ricerca. Fino a prima dei provvedimenti antielusione del 1992-1993 di Amato, l'aliquota IVA per le università era al 4 per cento. Chiediamo di riportarla allo stesso livello. Mi pare infatti intuitivo che se lo Stato dà 1.000 euro per espletare i compiti istituzionali di insegnamento e ricerca e poi ne reincamera immediatamente 200, si assiste a null'altro che a una partita di giro, rendendo poco più che simbolici i già scarsi finanziamenti. La seconda proposta riguarda l'IRAP. Attualmente le università hanno un'imposta imponibile IRAP assoggettata all'aliquota del 8,50 per cento, mentre per le imprese private grava solo per il 4,25 Con un trattamento privatistico dell'IRAP, il solo ateneo statale di Milano (che per il 2008 registra un esborso di 18 milioni di euro) conseguirebbe un risparmio di 9 milioni di euro. Le università, nel garantire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, rivestono un ruolo strategico per il Paese, non certo inferiore alle imprese produttive. Consideriamo quindi prioritario l'interesse delle università nel poter usufruire della riduzione dell'IRAP, al fine di sopperire alle carenze strutturali che da troppo tempo affliggono questo settore, di vitale importanza per il progresso e la competitività internazionale del Paese. Mi riferisco, in primo luogo, all'estrema precarietà del personale docente e ricercatore. L'abbassamento dell'aliquota creerebbe una fonte di risparmio non indifferente, tenuto conto dell'incidenza dell'8,5 per cento sul costo stipendiale del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, strutturato e non. I risparmi potrebbero essere utilizzati per la stabilizzazione di personale precario che svolge attività di didattica e di ricerca: docenti, ricercatori, dottorandi, specializzandi, assegnisti di ricerca, borsisti, contrattisti a tempo determinato eccetera. Chiedo, dunque, a chi ha a cuore l'istruzione universitaria di valutare questi interventi con la massima attenzione. *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, gli effetti della crisi finanziaria innescata lo scorso anno dal fallimento di numerose banche continuano a manifestarsi pesantemente sul sistema economico produttivo italiano, e non solo italiano. Tale crisi provoca una pesante recessione, che si è alimentata prima dalla paura e dalla sfiducia nei mercati finanziari, poi dalla caduta della domanda di beni e servizi, ed è stata causata prima dalla tensione sul mercato del risparmio, ora dalla caduta della domanda per l'aumento del tasso di disoccupazione.

(così come le recessioni dovrebbero essere affrontate), cioè con forti e massicci interventi di politica monetaria. In tal modo, si è frenata la valanga e apparentemente si è rimessa in moto, almeno nei grandi quadranti dell'economia mondiale, anche la domanda. Il clima di fiducia delle famiglie appare in miglioramento ed in misura molto minore anche quello delle imprese. È quindi passata la nottata? Cari colleghi, temo proprio di no, per tante ragioni che non ho qui il tempo di descrivere, ma che sono già state ben illustrate dalle relazioni di minoranza presentate ieri sera: la principale è che, a parte le politiche espansive, che consistono poi in produzione ed immissione di moneta, non è cambiato nulla sul piano della regolazione dei mercati finanziari; anzi, come avvertono numerosi osservatori, vi è il rischio che le condizioni che hanno determinato la crisi del 2008 si ripresentino potenziate per la massa di denaro che circola e per ciò che ne deriva. Infatti è quantomeno particolare che, pur in assenza di crescita della domanda, stiano aumentando in modo consistente tutti i prezzi delle materie prime, prime, non in relazione al naturale rapporto domanda‑offerta, ma alle aspettative che le stesse banche d'affari che hanno provocato la crisi del 2008 inducono nei mercati, con la conseguente accentuazione del rischio di nuove bolle finanziarie e nuovi tradimenti del mercato. La crisi non è alle spalle: temo anzi che nell'economia reale sia in gran parte davanti a noi. Infatti, quanto più l'economia finanziaria si distanzia da quella reale, tanto più si corrono rischi di ricadute ancor più gravi della malattia originaria.

Potrei confortare queste affermazioni con molti esempi, ma due provvedimenti ci dicono quanto le politiche governative abbiano battuto fuori tempo. L'anno scorso, la riduzione dei costi degli straordinari, mentre arrivava l'ondata della cassa integrazione guadagni, e la defiscalizzazione degli utili reinvestiti mentre scomparivano gli utili delle aziende: sono episodi sintomatici della non comprensione della natura recessiva di questa crisi. Eppure la crisi c'è, ed è pesantissima: nelle imprese dei settori manifatturieri si dichiarano cali di fatturato che per i settori di punta - lo sottolineo - vanno ben oltre il 50 che si trasformano in crisi di liquidità, di occupazione e, in prospettiva, in una grave crisi di competitività. Ad esserne coinvolte sono le imprese più dinamiche, che sviluppano investimenti e sono orientate all'alta specializzazione e all'*export*. La domanda di consumi ristagna, i risparmi delle famiglie si assottigliano ed il credito è molto problematico. A questa crisi non si può reagire con l'immobilità che finora ha caratterizzato l'azione di Governo: è il momento del coraggio riformatore, non della titubanza e dell'incertezza. È necessario sostenere la domanda, quindi vanno rimessi i soldi in tasca agli italiani e prima di tutto a quelli che ne hanno di meno. Va data certezza sul futuro occupazionale, con il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, da attuare non da solo, ma assieme alla riforma ed all'estensione degli stessi. Non mancano le proposte: confrontiamoci. È necessario far ripartire la leva della domanda pubblica, sbloccando anche attraverso una revisione del Patto di stabilità tutto quanto è finanziato e finanziabile a breve. Non mancano le proposte: confrontiamoci. Bisogna indurre comportamenti responsabili delle banche, oltre che verso i loro bilanci, anche verso l'economia. Anche qui non mancano le proposte; confrontiamoci. Bisogna utilizzare l'extragettito da scudo fiscale, la cui dimensione è ancora ignota, non per finanziare il bilancio corrente o una spesa pluriennale (sarebbe assurdo), ma per opere pubbliche necessarie e rapidamente cantierabili, per costruire infrastrutture moderne ed indispensabili per il Paese. Bisogna accelerare i pagamenti tra committenti e fornitori, a partire da quelli delle pubbliche amministrazioni. In questo senso, c'è stato qualcosa di molto colpevole da parte del Governo e dell'amministrazione dello Stato. L'efficienza della pubblica amministrazione, adesso, deve avere un indicatore che deve valere più degli altri: i termini e l'efficienza nei pagamenti, lo smaltimento dei residui passivi, la messa in campo di misure di controgaranzia pubbliche sui crediti che le imprese hanno maturato verso la pubblica amministrazione. È assurdo che una piccola impresa si veda negare finanziamenti da una banca perché non è ritenuto credibile il suo debitore, che è lo Stato o una pubblica amministrazione.

ma anche operando per modificare Basilea 2, svolgendo quindi un'azione internazionale. Bisogna trovare strumenti che canalizzino (con più fantasia e con un po' più di

È un delitto non rifinanziare il 55 per cento per le ristrutturazioni edilizie ed è un delitto perché lo si fa dicendo che è una legge che attira troppo; ciò vuol dire che è una legge che funziona.

suoi concorrenti irregolari. Si tratta di misure urgenti e indispensabili, ma prive di consistenza se non accompagnate da riforme strutturali che rendano credibile ai cittadini e ai mercati una reale volontà di cambiamento e di innovazione del nostro Paese. Concludo questo mio intervento, dicendo che ci sono cifre inconfutabili: c'è una crescita della spesa pubblica, c'è un aumento della pressione fiscale, c'è una crescita del costo della corruzione e dell'evasione fiscale (come dice la Corte dei conti), c'è una crescita dei disoccupati e c'è una caduta dei fatturati dei settori produttivi.

il premio Nobel Amartya Sen, solo la democrazia consente di correggere, quando ci sono, gli errori delle politiche economiche. Solo con il confronto e con la democrazia tali errori si possono, assieme, risolvere. *(Applausi

Per il 2010 viene infatti proposta una finanziaria snella, leggera, che si sostanzia in soli 3 articoli. Le norme contenute nel provvedimento in esame si limitano a fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio a disporre la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati, tenendo presente che il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente e il disegno di legge finanziaria hanno visto anticipati buona parte dei loro effetti dalle disposizioni previste dal decreto-legge n. 112 del 2008, con cui si è provveduto alla definizione dello scenario finanziario per il triennio 2009-2011, e dal decreto‑legge n. 78 del 2009, contenente misure anticrisi,

che devono ritornare ad essere al centro dell'azione del Governo. Il dibattito sulla questione meridionale ha fatto attentamente riflettere l'Esecutivo perché questa area del Paese registra un forte peggioramento delle condizioni economiche e sociali, con una programmazione insufficiente, che, purtroppo, ripete gli errori del passato. Oggi non possiamo più commettere gli stessi errori: occorre concentrare le risorse su obiettivi di carattere strategico che siano sviluppati anche come occasione per riqualificare gran parte della struttura economica nazionale. Questo tentativo, abbandonando ogni retorica, può e deve divenire concreto. Occorre, quindi, utilizzare al meglio i fondi a disposizione di questo progetto, che sono ancora ingenti nonostante i tagli effettuati. Le risorse destinate al Mezzogiorno ammontano a circa 60 miliardi di euro: esiste, quindi, la possibilità di utilizzare questo *budget*

e prevedere procedure di sostituzione in caso di inadempienza da parte degli enti locali. Su tale argomento è superare con la massima chiarezza i vecchi alibi e le vecchie diatribe, che ancora esistono, fra i diversi livelli istituzionali e, precisamente, fra Regioni e Stato centrale.

motivo, l'Italia del Sud ha bisogno innanzi tutto di una struttura bancaria autonoma legata ai propri territori. L'idea di una nuova Banca del Mezzogiorno non è

Signor Presidente, signori del Governo, colleghi senatori, il mio intervento sarà settoriale, limitato alla sanità e alla Protezione civile,

Noi speriamo che questa maggioranza, nel confronto con l'opposizione, abbia il coraggio di risolvere alcuni nodi illustrati durante il dibattito. Mi preme di nuovo confermare

dico sommariamente - riducendo le tasse sui salari, sul lavoro dipendente e sulle piccole imprese. Voi, invece, pensate di fare tutt'altra cosa. Noi pensiamo che la crisi debba servire per una riforma d'ordine generale della finanza pubblica e invece stiamo perdendo questa occasione. Del resto, abbiamo degli esempi in Europa: la Francia e la Germania stanno utilizzando il periodo della crisi per riformare l'intero sistema. Ci compiacciamo che quest'anno ci siano meno regalie dello scorso anno, perché lo scorso anno si è esagerato. Mi rivolgo soprattutto agli amici della Lega Nord, dai quali non accettiamo lezioni

Credo che dobbiamo avere un nuovo atteggiamento culturale durante la finanziaria, e soprattutto vi chiediamo più rispetto del Parlamento: questa è l'occasione per chiedere al Governo più rispetto per il Parlamento, come lo chiedono anche tante e tante componenti al vostro interno.

pochi lo avevano considerato. Noi abbiamo richiamato il Governo a sedersi al tavolo delle trattative con le Regioni. Il confronto è avvenuto, e credo che questa collaborazione istituzionale

Anche ieri il Presidente del Consiglio ha fatto intendere che uno degli obiettivi di questo Governo è quello di riordinare e riformare, a suo dire,

e lo Stato, il Governo e il Parlamento hanno l'obbligo di garantire l'erogazione di questo servizio, che deve essere uguale per tutti. Questa è la vera riforma che dobbiamo portare avanti nel settore della sanità, non creare barriere regionali, come sta avvenendo in alcune aree.

non riguarda la persona, ma si diventa poco credibili nei riguardi dei cittadini. Il commissariamento è un atto eccezionale e gravissimo nella Repubblica delle autonomie.

la sofferenza non si espone, non deve dare pubblicità, a chicchessia. Alla sofferenza si risponde con la soluzione dei problemi. Ecco perché diventa assurdo che, dopo lo *spot* pubblicitario del terremoto del Molise tramite il mio comune (dove - ripeto ancora una volta - sono morti 26 bambini e ora si sta trasformando in un bellissimo paese ricostruito), dopo sette

o almeno a quelli relativi alle quote di cofinanziamento, a carico degli enti locali, di opere decise dal CIPE. Abbiamo anche insistito sul fatto che per gli enti locali virtuosi, che si indebitano per fare investimenti,

modo esistono dei vincoli piuttosto stretti della finanza pubblica italiana che non consentono di prendere in esame l'insieme degli emendamenti da noi presentati. Il confronto con l'ANCI è sicuramente una realtà di fatto, ma se in questo ramo del Parlamento, dove si esamina la finanziaria, il Governo e la maggioranza diranno di no agli emendamenti da noi presentati, anche a quelli meno costosi e meno impegnativi, questo sarà in ogni caso un pessimo modo per avviare un confronto. Poiché sappiamo che anche la maggioranza

Durante la discussione è stato affermato che vi sono già alcune modifiche intervenute sul patto di stabilità interno per il 2009 e che ciò non consentirebbe ulteriori interventi.

Ma dette misure sono del tutto insufficienti, poiché hanno liberato solo 1,8 miliardi di euro circa, a fronte di ben 44 miliardi bloccati dalla normativa vigente. Deve essere chiaro cosa sta succedendo. Il patto di stabilità interno interviene sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione e su quello degli enti locali ponendo dei vincoli all'utilizzo delle risorse che Comuni e Province hanno disponibili, in cassa; esso induce la creazione di residui passivi ed impedisce, ad esempio, il pagamento anche di stati di avanzamento di opere già appaltate. Per tali motivi c'è una fortissima preoccupazione, un vero e proprio allarme da parte di tutte le categorie economiche, l'ANCE in primo luogo (ma non solo), e delle organizzazioni sindacali. È evidente che, in una fase di difficoltà economica e di crisi occupazionale come l'attuale,

spesa per investimenti di questo Paese sia promossa dai livelli territoriali, e in una fase di crisi sarebbe estremamente necessario consentire a questa leva di agire. Per gli anni a venire, tra l'altro, il patto di stabilità interno prevede restrizioni ulteriori. In modo particolare, nel triennio 2009-2011 è richiesto, in termini di miglioramento dei saldi, un contributo pari a ben 4 miliardi e 145 milioni di euro. è emerso un altro elemento di discussione con il vice ministro Vegas in merito ad alcuni dati. Ora, quando si mettono a confronto i dati sull'indebitamento netto dei vari comparti della pubblica amministrazione, lo si fa evidentemente

anche l'ANCI nei documenti presentati, avvengono in modo omogeneo e non considerano il peso del debito pubblico. Sono fatte in modo da consentire delle comparazioni omogenee.

Ancora, l'indebitamento netto della pubblica amministrazione nel suo complesso - e qui cito un dato ISTAT del 22 ottobre - nel 2008 è aumentato di 19,8 miliardi di euro.

si prende in considerazione l'andamento dell'indebitamento netto e dunque della stessa grandezza per quanto riguarda i Comuni, si

È la conferma di un *trend* di lungo periodo che, a partire dal 2004, ha determinato un miglioramento del saldo di bilancio dei Comuni di oltre 2,5 miliardi di euro, mentre nello stesso periodo il miglioramento della pubblica amministrazione è stato di 5,6 miliardi di euro. Ciò vuol dire che quasi la metà del miglioramento è avvenuto a carico dei Comuni. Questo a significare che è del tutto sproporzionato il peso che i Comuni hanno avuto sul miglioramento dei saldi pubblici rispetto al loro peso sulla spesa complessiva della pubblica amministrazione. In altri termini, mentre la spesa dei Ministeri centrali è evidentemente fuori da ogni controllo, la spesa dei Comuni è invece messa sotto controllo ma in modo eccessivo, tale da produrre effetti depressivi sull'insieme dell'economia. Ricordo ancora - e concludo, Presidente - i dati relativi all'ICI. Non è stato interamente restituito il mancato gettito per la perdita dell'ICI sull'abitazione principale ai Comuni. Si evidenzia inoltre ancora una riduzione dei trasferimenti di 200 milioni di euro per il 2010, che i cosiddetti costi della politica fanno sì che vi siano altre centinaia di milioni di euro che mancano alle casse dei Comuni. In considerazione di una questione fondamentale, sulla quale il nostro Gruppo continuerà ad insistere con forza nel corso della discussione, nella certezza che anche ampi settori della maggioranza la pensino

di ottenere risultati importanti sul piano della tenuta della finanza pubblica, che ha permesso al nostro Paese di mantenersi entro un quadro di stabilità e di credibilità nel contesto mondiale, in una difficilissima situazione di crisi, in cui i nostri indicatori si sono modificati in linea con le variazioni all'interno del quadro europeo. Così, la previsione sui nostri indicatori economici, per quest'anno e per gli anni prossimi, è sostanzialmente in linea - cosa non usuale - con gli indicatori dei maggiori Paesi

parte nostra avevamo il forte vincolo del grande indebitamento, una leva su cui il nostro Paese non può e non poteva agire perché il nostro indebitamento è già a livelli molto superiori di quelli cui pensa di arrivare la maggior parte dei Paesi europei alla fine di questo percorso di crisi, di aiuto e sostegno all'economia. In un quadro siffatto non si può che apprezzare la politica

nel quadro del mantenimento dei conti pubblici, di cominciare ad adottare politiche di sviluppo ed espansive.

della nostra parte politica da ben prima che venissero evidenziati dal centrosinistra: la riduzione delle tasse per le imprese e le famiglie, la spesa per gli investimenti, la spesa per la sicurezza, la spesa per l'istruzione e l'università. Sono temi rispetto a cui la nostra coalizione è nata e si è cementata, fanno parte del nostro DNA politico, e non vedo come ci si possa meravigliare che

normale e giusto che il Parlamento e i parlamentari siano sensibilizzati dall'opinione pubblica e dal territorio su alcune tematiche e alcuni bisogni di cui naturalmente essi devono farsi carico. Credo che il lavoro parlamentare svolto sia stato positivo

i senatori Saia e Latronico, che hanno tenuto sempre alto il livello della discussione a cui - devo ammettere - anche l'opposizione ha partecipato in termini positivi e costruttivi, offrendo un contributo di idee. È un dibattito

poco fa si parlava, è vero che sono tanti gli sprechi, è vero che buona parte delle Regioni del Sud è oggi sotto commissariamento, ma è vero anche che il nostro livello di spesa sanitaria è inferiore a quello degli altri Paesi europei,

che la domanda è crescente per quanto riguarda lo svilupparsi delle tecnologie in campo sanitario e rispetto all'invecchiamento della popolazione e all'arrivo di qualche centinaia di migliaia di immigrati, i quali hanno e costituiscono anch'essi domanda sanitaria. L'azione del Governo si è concentrata e si sta concentrando, secondo me opportunamente, sulla partita degli ammortizzatori sociali. È vero che oggi vi sono buoni margini rispetto alla domanda esistente, ma non bisogna abbassare la guardia perché nessuno di noi può prevedere gli effetti

il percorso che il Governo ha delineato e che la maggioranza sta portando avanti, sempre mantenendo alto il livello del dibattito sulle ulteriori misure che possono essere introdotte attraverso il percorso parlamentare.

del dibattito parlamentare di questi giorni. La partita del sisma dell'Abruzzo - come già qualcuno ha detto

alla possibilità di ottenere risorse attraverso gli strumenti messi in campo dal Governo, sul fatto che quelle risorse non ci fossero, non ci fosse copertura finanziaria, non fosse possibile erogarle. Credo che a sei mesi dal sisma

Oggi c'è da gestire la fase delicata della ricostruzione pubblica delle infrastrutture, dei centri storici. La stiamo affrontando, ma anche per tale fine ci sono delle risorse, come ha chiarito il CIPE qualche settimana fa. Credo che anche in questa partita il Governo abbia dato un esempio

Signor Presidente, onorevoli colleghi, da quando è iniziata la crisi economico-finanziaria, che ha investito il complesso dei Paesi industrializzati, l'Esecutivo ha alternato, di volta in volta, prese di posizione assolute dimostratesi sempre in antitesi con quella che era la realtà dei fatti. Citando un famoso regista italiano potrei dire che: chi parla male, pensa male e, aggiungo, In questi mesi siamo passati inizialmente dalla negazione della crisi (mentre tutti i Governi del mondo assumevano iniziative capaci di far fronte ad essa), alla sua sostanziale sottovalutazione (con una politica dilatoria, sperando che il malato guarisse da solo), alla sorprendente fine della crisi. Una commedia in tre atti che neanche i più grandi commediografi avrebbero potuto ipotizzare. Ma, come purtroppo ben sappiamo, la commedia spesso si trasforma in tragedia. La realtà che viviamo oggi nel nostro Paese si avvicina molto alla tragedia: centinaia di migliaia di lavoratori in cassa integrazione che vivono con l'angoscia di non veder rinnovata la cassa integrazione nei prossimi mesi e di non rientrare in azienda; centinaia di migliaia di lavoratori precari che per primi sono stati esclusi dai cicli produttivi e che non hanno alcuna protezione sociale; i tanti precari della scuola che vivono con crescente angoscia il loro futuro occupazionale; i milioni di nostri connazionali che vivono (o sopravvivono) sotto la soglia della povertà; le migliaia di piccole e medie imprese che rischiano di chiudere i battenti anche a causa della stretta creditizia in atto in Italia. A questa realtà, non fatta di fredde statistiche, ma di uomini e donne, la legge finanziaria, di cui oggi proseguiamo l'esame, non dà risposte. Una norma ragionieristica, svuotata da ogni strumento di politica di sviluppo e prigioniera delle beghe di maggioranza, discussa in stanze private e di cui ancora non ci è dato sapere il reale impianto finale. Ma nonostante il nostro giudizio fortemente critico su questa manovra, in relazione alla mancanza di misure a sostegno del potere d'acquisto del redditi dei lavoratori e dei pensionati, a sostegno della domanda interna, in relazione all'inesistenza di strumenti di protezione sociale e per il contrasto alla povertà, abbiamo messo in campo proposte emendative ed ordini del giorno che intervengono in questi settori e che, se assunte dalla maggioranza, potrebbero dare risposte all'emergenza sociale in atto nel nostro Paese. Come abbiamo già avuto modo di evidenziare durante la discussione in Commissione lavoro, riteniamo indispensabile l'assunzione immediata di alcuni strumenti inderogabili. Penso in particolare alla ridefinizione ed estensione su base universalistica del sistema degli ammortizzatori sociali, dando piena ed immediata attuazione alla delega conferita in materia al Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 28 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, all'adozione di interventi di defiscalizzazione dei redditi da lavoro dipendente e da pensione, anche dando seguito a quanto previsto dal Protocollo sul *Welfare* del 23 luglio 2007, allo scopo di produrre effetti immediati sulla ripresa del potere d'acquisto dei medesimi; al ripristino della dotazione economica e l'ulteriore incremento del Fondo per le politiche sociali, prioritario strumento di contrasto alle emergenze sociali e per l'implementazione di politiche sociali attive e di attuazione dei diritti di cittadinanza che, al contrario, viene ulteriormente ridotto rispetto a quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2009. Riteniamo inoltre necessario prevedere, in conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, lo stanziamento occorrente per il raddoppio della cassa integrazione ordinaria come richiesto da tempo dal complesso delle organizzazioni sindacali - dalle attuali 52 settimane alle 104 settimane. Voglio poi richiamare l'esigenza di stanziare risorse adeguate e strutturali per il rinnovo triennale dei contratti del pubblico impiego, attuare anche misure di carattere finanziario per dare una risposta ai precari che ci sono in questo settore. un complesso di proposte migliorative, insieme alle molte altre che illustreranno i miei colleghi, che danno il senso della serietà con cui approcciamo questa discussione, e che richiederebbero pari serietà da parte della maggioranza.

Paese? Bisogna investire le risorse che si possono reperire anche dal cosiddetto scudo fiscale per sostenere con misure immediate il potere di acquisto di salari e pensioni. Si tratta di fare una scelta chiara: chiedo alla maggioranza di utilizzare queste risorse per una misura di carattere straordinario volta alla defiscalizzazione della tredicesima mensilità dei lavoratori dipendenti e dei pensionati con redditi medio-bassi. Qui sta la priorità. È indispensabile sostenere il reddito e rilanciare i consumi. Si tratta di una misura che il Governo potrebbe assumere nell'immediato, anche con lo strumento della decretazione d'urgenza, visto che ne fa uso continuo. Abbiamo bisogno di discutere, di avere messaggi chiari e di dare risposte alle persone che più sono a disagio in questo Paese. Abbiamo bisogno di dare una risposta forte

Per questo vogliamo dal Governo una risposta chiara e precisa. Non vogliamo un "quarto tempo" e che dopo tutte le promesse, le sottovalutazioni, gli errori a questo punto ci sia la beffa della mancanza di risposte al Paese, che rischia di arretrare sempre di più.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, nella manovra finanziaria al nostro esame il Governo conferma nuovamente che le dichiarazioni di intenti non sono state trasformate in concreto in misure di indirizzo e di sostegno alle famiglie ed all'economia. Si tratta di un documento privo di contenuti significativi e dunque lo reputo inadeguato a rispondere alle difficoltà economiche e finanziarie che coinvolgono l'intero Paese. Mancano totalmente misure forti e incisive a favore delle famiglie ed ancora una volta non sono state messe a disposizione adeguate risorse finanziare, in particolare in merito alla disponibilità del credito per le piccole e medie imprese. La caduta del PIL registratasi nell'anno in corso ha avuto un pesante impatto occupazionale e senza misure di incentivazione a favore delle imprese non sarà possibile riassorbire la forza lavoro lavoro inutilizzata. Particolarmente grave è che si prevedono soprattutto licenziamenti di lavoratori di mezza età la cui ricollocazione sul mercato del lavoro sarà molto ardua. A tale riguardo, è necessaria la predisposizione di una riforma organica del sistema degli ammortizzatori sociali unitamente a misure fiscali, quali la deduzione della componente lavoro dalla base imponibile dell'IRAP. Da questo Governo, che tanto parla e poco concretizza, mi sarei aspettato di più. Saluto con favore una politica di rigore dei conti pubblici; tuttavia si potevano e si dovevano effettuare dei tagli alla spesa pubblica inefficiente. Non possiamo prescindere dal predisporre riforme strutturali senza le quali questo Paese non potrà tornare a crescere. C'è bisogno di una svolta. Sollecito nuovamente il Governo ad adottare misure concrete per lo sviluppo del sistema turistico in considerazione del crollo verticale registratosi questo anno per quanto riguarda l'afflusso in Italia di turisti stranieri. stranieri. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i casinò proposti dal Ministro per il turismo non sono certamente la risposta giusta. Sarebbe, invece, utile prendere a modello l'iniziativa dei Governi francese e tedesco, che hanno drasticamente ridotto l'aliquota IVA applicabile ai servizi turistici, portandola rispettivamente al 5,5 e al 7 per cento, rispetto al 10 per cento dell'Italia. Mi preme, a tal riguardo, ricordare che in Italia il settore del turismo, pur avendo uno dei maggiori potenziali, ha da tempo perso il suo primato storico nel mondo. Se il Governo non si decide ad adottare misure assolutamente necessarie per rimanere competitivi, come ad esempio il citato abbassamento dell'IVA, il tanto evocato rilancio del turismo resterà lettera morta. Appare particolarmente urgente risolvere alcune emergenze del nostro settore produttivo. Al riguardo, mi riferisco alla necessità di prevedere l'innalzamento del limite di deducibilità degli interessi passivi e a una diversa procedura per garantire una soluzione alle problematiche dei pagamenti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese creditrici, nonché alla mancata attuazione dell'IVA per cassa. Anche la mancata proroga degli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici agli anni 2011 e 2012 è semplicemente inaccettabile. La detrazione IRPEF del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica degli edifici andava potenziata in quanto ha dato risultati fortemente positivi sia in termini ambientali che economici contribuendo al rispetto dei parametri europei nell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra. Era una misura di impulso all'utilizzo delle fonti rinnovabili ed assolutamente necessaria per il sistema produttivo e occupazionale in una fase di grave recessione economica. Inaccettabile è altresì il fatto che non compaiano le consuete proroghe del settore agricolo, tra le quali cito il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, le agevolazioni contributive per le zone svantaggiate e montane, l'accisa zero per il gasolio utilizzato nelle colture in serra e le agevolazioni fiscali per la formazione della proprietà contadina. Nel corso di un'audizione il presidente della Confagricoltura, Federico Vecchioni, ha indicato gli interventi necessari per l'agricoltura, chiedendo espressamente di inserirli nella finanziaria 2010. Si tratta di circa 1,3 miliardi di euro, il cui finanziamento per 1,2 miliardi può essere garantito dai residui

negli ultimi anni ha subito pesanti tagli a scapito del Fondo di solidarietà nonché delle politiche di sviluppo e oggi, anche alla luce della forte crisi economica, versa in condizioni critiche. Non bastano interventi *una tantum*, ma dobbiamo dare segnali nuovi, attivando adeguate politiche di investimento, scommettendo sulla capacità di successo dei

che accanto a questi interventi necessari occorre urgentemente agire per l'alleggerimento della burocrazia, che grava pesantemente sulle piccole e medie imprese, già fortemente colpite dalla crisi. *(Applausi dai

noi dell'Italia dei Valori dobbiamo e vogliamo essere chiari sino in fondo: oggi stiamo discutendo di una finanziaria che non c'è, di un provvedimento del tutto inadeguato e insufficiente, che fa semplicemente da ponte tra ciò che non si è voluto fare prima e ciò che non si sa o non si vuole fare dopo. La verità, per dirla in tutta la sua interezza, è che la vera manovra finanziaria sarà quella che vedremo nei prossimi anni (se tutto va bene, nei prossimi tre). Quel poco che c'è ora non è altro che una sommatoria di contraddizioni, di altalene, di dati congiunturali e di eclatanti paradossi. L'hanno già detto tutti, per cui non intendo ripetere che il quadro dei conti pubblici è decisamente oscuro e prevede per fine anno un deficit pari al 5,3 e un debito al 115 per cento del PIL, con un fabbisogno dello Stato che è arrivato ad un incremento di circa 30 miliardi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La situazione dell'economia reale comincia ad essere oggetto di grave preoccupazione anche da parte di chi non può essere iscritto di comodo alla categoria dei catastrofisti. È di qualche giorno fa la notizia che l'amministratore delegato di Intesa San Paolo ha dovuto confermare che vi sono 250.000 imprese italiane a rischio di sopravvivenza. Il primo dato paradossale, allora, in questa finanziaria è che la manovra triennale avviata dal Governo nell'estate 2008, all'insegna della stabilizzazione dei conti pubblici, ci ha portato comunque in una nuova procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo. Certo, il ministro Tremonti ci ha detto che siamo in buona compagnia, visto che sono 20 gli Stati membri che non hanno rispettato le regole comunitarie. Certo, molte delle responsabilità vanno addebitate alla crisi internazionale, ma quando si è guardato con un'autoreferenzialità ossessiva e paranoica al bilancio e ai vincoli europei e si è pensato, come si è fatto, poco o nulla a curare i veri mali della nostra economia, le responsabilità appartengono anche alla palese volontà o incapacità del Governo di non adeguare la manovra triennale agli effetti della crisi stessa, facendo finta per troppo tempo che questa quasi non ci fosse. Anche ora, di fronte all'evidenza dei dati, al Paese viene ripetuto - come ha fatto sino a pochi giorni fa il Capo del Governo - che i conti pubblici sono rimasti sotto controllo può stare tranquilli, perché quando l'economia finalmente ripartirà, saremo in grado di rientrare dal disavanzo senza bisogno di manovre correttive, ma anche questo è falso. L'Europa ci dice che dovremo aggiustare il bilancio di un punto strutturale per i prossimi tre o quattro anni e questo significa circa 15 miliardi annui di tagli di spesa oppure di nuove tasse. Bisogna avere l'onestà di riconoscere che la crisi c'entra, ma fino ad un certo punto, e che il Paese, nonostante l'assenza colposa di necessari interventi anticiclici, si sta avviando verso un nuovo ciclo di aumento incontrollato della spesa primaria, simile a quanto già visto dagli italiani nel precedente Governo Berlusconi tra il 2001 e il 2006. I numeri di oggi ci dicono che la scelta messa in campo con il decreto-legge n. 112 del 2008 e basata su una logica prevalentemente di tagli lineari non solo non ha prodotto i risultati attesi, ma al contrario, rispetto alle previsioni, la stima delle spese al netto degli interessi sale a circa 25 miliardi. nello scarto di 11 miliardi, solo 3,7 miliardi sono i fondi per interventi anticrisi, come i pochi ammortizzatori sociali per i più fortunati, un *bonus* famiglia *una tantum*, la carta della povertà di 40 euro mensili. Il secondo dato paradossale, signor Presidente, è che, nonostante questa crisi sia stata definita, a ragione, la peggiore dal dopoguerra, questo Governo di fatto non ha preso finora decisioni significative di finanza pubblica. Un dato che, insieme ad altri, deve farci riflettere è lo studio dell'ISAE, secondo il quale l'insieme degli Stati membri dell'Europa ha disposto provvedimenti anticrisi per un totale pari all'1,1 per cento del PIL nel 2009 e allo 0,7 per cento Per l'Italia, invece, il totale di misure di stimolo fiscale per il 2009 e per il 2010, comprensivo di misure dirette alle famiglie, al lavoro e alle imprese, è pari allo 0,0. Ma per noi dell'Italia dei Valori non è questo il problema; o almeno non è solo questo, perché non pensiamo che dalla crisi si esca con lo "zero virgola". Vorrei invece che riflettessimo anche su un altro dato, frutto dello studio di organismi imparziali: se l'Italia dovesse uscire dalla recessione, a bocce ferme (come sta facendo il Governo) e crescendo con lo stesso ritmo con cui è cresciuta nei dieci anni che hanno preceduto la crisi, ci vorrebbero ben 15 anni per recuperare il terreno perduto. E terreno perduto significa persone senza lavoro, famiglie in povertà alimentare, disuguaglianze sociali. Non possiamo perciò permetterci di continuare a guardare alla finestra, senza affrontare i problemi strutturali dell'economia italiana. Un esempio tra gli altri: in Italia il 95 per cento delle aziende ha meno di dieci addetti ed è quindi soprattutto da queste piccole imprese, che danno lavoro a quasi un italiano su due, che ci dobbiamo aspettare il maggiore contributo al rilancio della nostra economia. E se i piccoli imprenditori stanno male, i lavoratori delle piccole imprese stanno ancora peggio. Eppure i nostri ammortizzatori sociali, i migliori del mondo (come li ha definiti Brunetta), li trattano peggio dei lavoratori delle grandi imprese. Chi ha la fortuna di avere un contratto a tempo indeterminato riceverà un assegno di 600 euro per 8 mesi, mentre sono più di un milione e mezzo i lavoratori senza alcuna tutela e un altro milione quelli che possono accedere solo ai sussidi a requisiti ridotti. Il terzo elemento paradossale è che, nonostante gli sforzi propagandistici del Governo, questa finanziaria non riesce a convincere proprio nessuno, soprattutto non piace a nessuno. Non piace ai Comuni, che nel confronto con il totale della pubblica amministrazione hanno fatto ampiamente la loro parte, hanno già dato, visto che il loro contributo al contenimento del disavanzo di bilancio è stato il maggiore sul totale delle amministrazioni pubbliche, e che per raggiungere questi risultati, dopo aver tagliato sulle prestazioni sociali, hanno dovuto sacrificare una parte cospicua della spesa per investimenti. Per i Comuni la situazione è drammatica. Tra le minori entrate dovute all'abolizione dell'ICI sulla prima casa, il taglio dei trasferimenti erariali relativi ai fabbricati ex rurali, il taglio per i risparmi sui costi della politica e la riduzione di 200 milioni di euro del fondo ordinario, per il 2009 l'importo delle minori entrate sale a un miliardo e 220 milioni di euro, mentre per il 2010 la perdita per i Comuni è stimata pari a un miliardo e 350 milioni di euro. Sul patto di stabilità - lo ha ricordato il collega Vitali - non è servito a nulla il decreto legge n. 5 del 2009, che dispone l'esclusione dal patto di alcuni tipi di spesa solo per quei Comuni che presentano determinati requisiti e per un importo non superiore a quello autorizzato dalla Regione di appartenenza. L'intervento è stato adottato soltanto in due Regioni. A poco è servita l'ultima modifica apportata con il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che ha permesso agli enti locali di utilizzare un importo pari al 4 per cento dei residui passivi accumulati al 2007, perché anche questa misura è risultata insufficiente,

più disposti al dialogo, perché ormai anche loro lamentano che la cautela imposta dai conti pubblici non basta più a giustificare l'esigua quantità di risorse messe in atto contro la crisi che stiamo attraversando. Un rallentamento della recessione - mi rivolgo a chi se ne fa quasi vanto - non induce di per sé una ripresa dell'occupazione! Le stime OCSE prevedono una crescita del tasso di disoccupazione a due cifre, comportando la perdita di oltre 1 milione di posti di lavoro; non è più comprensibile, quindi, per il Paese perseverare in una strategia che si affida al meccanismo delle *una tantum*, assumendo il debito pubblico come alibi di un rigido vincolo di bilancio rispetto alla possibilità alternativa di politiche espansive. I sindacati ricordano che il Governo, sul sistema degli ammortizzatori sociali, in seguito all'accordo del febbraio scorso con le Regioni, aveva assunto un impegno e aveva fornito precisa assicurazione che sarebbe stato pronto a trovare risorse aggiuntive per le necessità future. Questa finanziaria non piace neppure - e il che è tutto dire - alla Confindustria che ha denunciato come il Mezzogiorno non possieda, nell'attuale drammatico momento di crisi, alcuno strumento attivo a livello nazionale per sostenere gli investimenti delle imprese. In particolare, il credito di imposta per gli investimenti - il cosiddetto *click day* - ha esaurito già a settembre 2008 l'intero stanziamento fino al 2015 e nulla fa prevedere a legislazione vigente che le risorse che si dovessero liberare potranno essere impiegate per anticipare la fruizione del credito e per estendere la platea dei beneficiari. beneficiari. Questa finanziaria non piace alle associazioni di categoria, artigiani, commercianti, esercenti, che chiedono di fare di più perché, se è vero che non ci sono scorciatoie, è altrettanto vero che non ci sono alternative: più crescita e più reddito richiedono più produttività e minore carico fiscale. Le riforme strutturali richiedono tempi lunghi e consensi ampi, ma alcuni provvedimenti possono e devono essere adottati fin da subito in una possibile compatibilità con una strategia di finanza pubblica. Questa finanziaria non convince - e anche qui è tutto dire - neppure l'Associazione nazionale costruttori edili, perché dal disegno di legge emerge una riduzione delle risorse per investimenti e nuove infrastrutture di oltre il 7 per cento in termini reali rispetto all'anno precedente. Non è solo un problema di stanziamenti, ma è anche e soprattutto un'esigenza di accelerazione della spesa per investimenti. Il tempo, in momenti del genere, è decisivo ed è necessario accelerare l'effettivo avvio del piano delle infrastrutture prioritarie, che per noi non significa il ponte di Messina, ma attuazione particolare per i programmi di opere medio-piccole di pronta cantierizzazione, interventi di edilizia scolastica e carceraria e quelli per l'emergenza Abruzzo che, oltre a rispondere ad esigenze specifiche, possono dare un sostegno immediato a comparti diffusi della nostra economia. Questa finanziaria non convince neppure la Corte dei conti, che ha evidenziato un aspetto meritevole, signor Vice Ministro, di un'attenta considerazione, perché ancora una volta per noi il Governo sta sbagliando e sarebbe un'ulteriore recidiva. Ponendo infatti a confronto le nuove stime governative, le previsioni ipotizzano,

In altri termini, il Governo ritiene che l'uscita dalla recessione si tradurrà nel medio periodo in un innalzamento della crescita dell'economia italiana di quasi mezzo punto all'anno, in ragione di un automatismo di una ripresa del commercio internazionale e di un effetto rimbalzo dell'economia. È quello che la Corte dei conti chiama «facile ottimismo», come risulta dai verbali dell'audizione in Commissione bilancio. Per noi, sostanzialmente, è continuare a dare numeri sulla pelle degli italiani. In ultimo, ma non da ultimo, un'altra considerazione: le polemiche di questi giorni dentro Governo e maggioranza dimostrano che questa finanziaria non convince neppure chi la dovrebbe votare. Una cosa, almeno, ci avete aiutato a capire rispetto a quanto noi da tempo stiamo dicendo: era e rimane strumentale una lettura della situazione nel nostro Paese fondata sulla contrapposizione tra un partito del rigore, impersonato dal Ministro dell'economia, e un partito della spesa, rappresentato da chi si permette, per lesa maestà, di contestare la politica di Tremonti. A parte che per noi resta difficile e poco credibile assegnare la medaglia del rigore contabile a un Ministro che, dopo aver dichiarato la messa in sicurezza del bilancio, si trova ora dinanzi ad un deficit del 5 per cento e a A parte che, primo fra tutti, a dare un brutto esempio del partito della spesa è proprio il Presidente del Consiglio con il suo, come al solito, improvvisato ed elettoralistico annuncio del taglio dell'IRAP senza la più pallida indicazione del come coprire il conseguente fabbisogno dei conti pubblici. A parte emendamenti della maggioranza che fantasticano di riduzioni immediate di 20 miliardi della spesa per acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche e di tagli di 15 miliardi di trasferimenti a fondo perduto alle imprese, senza tenere conto che in Italia di riduzioni dei cosiddetti consumi intermedi sono piene le storie di molte finanziarie e che poi si è visto che le spese immancabilmente rimbalzavano l'anno dopo. A parte tutto questo, con questa questo, con questa finanziaria, ancora una volta, il Governo ha avuto l'irresponsabilità di trasformare il presunto rigore in una dannosa immobilità e, nella situazione in cui si trova il nostro Paese, questo significa ancora una volta voler abdicare al compito di governare operando le scelte prioritarie rispetto alla soluzione dei problemi prioritari. apre una nuova finestra"). Onorevoli colleghi, previe intese intercorse tra i Gruppi, comunico che la seduta di oggi pomeriggio è anticipata alle ore 16 e potrà concludersi anche oltre le ore 20,30, al fine di completare, entro questa sera, le votazioni degli emendamenti al disegno di legge di bilancio.